a pochi metri da qua, oggi inizierà a ricevere un ultimo saluto. È difficile trovare le parole adeguate per affrontare una straordinaria una straordinaria montagna, una vetta del cinema italiano. Qualcuno, citando un suo film, l'ha definito l'ultimo imperatore del cinema, ma credo che non gli sarebbe piaciuta la parola «ultimo»:

un grande maestro, un grande genio, che la nostra creatività e la nostra storia devono essere ancora capaci di far emergere. Ecco, la storia di Bertolucci interseca straordinariamente quella del nostro Paese: egli era così tanto italiano

Grazie,

È più difficile sognare guardando fuori e incontrando il mondo, però però c'è una chiamata alla partecipazione civile. E quella chiamata è tutta dentro quello che probabilmente è il suo grande capolavoro, «Novecento», il film che davvero ha raccontato, meglio di qualsiasi saggio, che cosa è stato non il Novecento italiano, non il Novecento europeo, ma tutto il Novecento: la scoperta del popolo, l'ingresso del popolo nella storia, la capacità delle masse popolari di diventare nazione, di diventare partecipi e di affrontare questo con tutte le contraddizioni, con le contraddizioni degli scontri, con le contraddizioni della violenza, senza mai perdere - perché questa era una delle grandezze di Bertolucci - la singolarità di ogni vita. C'era l'individuo, c'era la persona, senza che ci fosse l'individualismo, senza perdere l'idea che l'individuo è sempre inserito dentro a un contesto sociale e a un contesto di relazioni. Ecco, io credo che in sedici Grazie,

la sfida della relazione tra l'uomo e la donna. È un'idea di protagonismo femminile che era assolutamente presente nelle corde di quel tempo. Ecco, Bertolucci ha attraversato tutto questo e lo ha saputo fare perché ha sempre tenuto le antenne alzate sul mondo, ha sempre saputo incrociarsi con le altre arti e ha sempre saputo ascoltare i differenti stimoli che venivano anche dalla modernità. Proprio in quel film, pensiamo a come egli innovi la tecnica e innovi anche dal punto di vista musicale. Però ha saputo essere sempre nazional-popolare, parlare a chiunque: alle persone colte, che potevano magari cogliere la raffinatezza della sua citazione, ma anche all'uomo semplice, alla donna del donna del mercato, alla donna del bar, ed emozionarla, perché questa è la grandezza dell'arte, la grandezza della verità assoluta dell'arte, una verità individuale che tocca le corde di ognuno di noi che ci fa riconoscere dentro quel grande schermo. Ecco, le parole non possono raccontare tutto questo. Sarebbe bello che, in questo momento, in quest'Aula potessero trascorrere veramente delle immagini. Vorrei concludere il mio intervento così, signor Presidente, con un richiamo a tutti noi. Questa è un'Aula in cui tante volte ci scontriamo, in cui qualche volta viviamo ed esercitiamo anche le miserie; esercitiamo il potere con tutte le sue contraddizioni. Noi dobbiamo sempre avere il coraggio di guardare alto, di guardare lontano; la grandezza degli artisti ci stimola proprio a questo. Ogni tanto, uscendo da quest'Aula, prendendo in mano un libro o guardando un film straordinario - e magari in questi giorni tornando a guardare uno di quei grandissimi film di Bernardo Bertolucci

Signor Presidente, anche il MoVimento 5 Stelle esprime il cordoglio per la scomparsa di un grande maestro come Bernardo Bertolucci. Io userò poche parole; tra l'altro, questa è un'Assemblea un po' distratta per una commemorazione, mi si consenta almeno questo. Userò poche parole perché, per chi ama il cinema, per chi ha tentato di farlo, per chi semplicemente si trova anche per caso a farlo, figure come quella di Bernardo Bertolucci sono un punto di riferimento: appartengono alla storia del nostro Paese, non solo alla storia del cinema, ma alla storia culturale, alla storia migliore di questa Italia, Italia, che tra l'altro ha guadagnato notorietà nel mondo. È inutile che ricordi che i film di Bernardo Bertolucci sono considerati una delle espressioni più alte, più complesse e più compiute dell'arte cinematografica italiana.

per lo stesso Pasolini, quando si presentò senza praticamente nulla e iniziò a Roma il suo percorso cinematografico. Io però vorrei anche sottolineare come la scomparsa di artisti come Bernardo Bertolucci sia non solo una perdita culturale enorme ma che abbia anche un risvolto, se vogliamo, pratico, concreto, ovvero il fatto

di suo immette nella propria opera. Quindi il discorso è ricco e complesso, tra l'altro esteticamente assolutamente di pregio (pensate al sodalizio con Vittorio Storaro). Insomma Insomma è importante perché non avere più quello sguardo sulla realtà, non avere più quel punto di riferimento oltre a rattristarci, in qualche modo ci disorienta.

Grazie,

Bertolucci ha rappresentato, nella sua lunga carriera, la grande evoluzione del cinema italiano. Quel cinema che è diventato grande per il suo modo di guardare il mondo, la realtà. In molti suoi film vi è anche un un connubio con il mondo della letteratura che molto spesso - penso a «Il conformista» - ha fatto rivivere,

che hanno dato lustro non soltanto alla poesia, alla letteratura e al cinema ma che hanno dato una possibilità di vicinanza e di reinterpretazione

come Paese, per aver avuto un grande maestro come Bertolucci.

tra comunismo e fascismo, su momenti di grande passaggio. Quelli appena citati sono solo alcuni dei grandiosi successi di quello che è stato comunque un figlio della nostra Italia. Bertolucci ha dato lustro alla Nazione, vincendo qualsiasi premio, compresi un Oscar come migliore regista e un Leone d'oro alla carriera al Festival del cinema di Venezia. Quindi, come dicevamo, egli lascia un grande vuoto nei suoi familiari, ma anche in noi, che abbiamo avuto il privilegio di essere spettatori dei suoi film. Diciamo addio a questo grande maestro e continueremo a seguire la sua arte, che invece resterà scolpita in eterno, attraverso i suoi film.

con le misure contenute nel decreto-legge in esame veniamo incontro alle esigenze delle persone che si sono trovate in difficoltà a causa della crisi economica e della pressione insostenibile del nostro sistema tributario. Non parliamo dei grandi evasori, esclusi da questo provvedimento, ma di quei contribuenti che non sono stati in grado di pagare le tasse per una situazione economica oggettivamente penalizzante. Veniamo inoltre incontro alle imprese, in particolare alle piccole imprese, introducendo misure finalizzate a ristabilire un nuovo rapporto di fiducia tra fisco e contribuente quale necessaria premessa per l'avvio di un graduale processo di riduzione della pressione fiscale e di semplificazione del sistema impositivo. in esame diamo quindi un segnale a quel nuovo ceto sociale debole e ai nuovi poveri, che i Governi precedenti spesso non hanno saputo riconoscere. Vogliamo quindi invertire il paradigma e volgere lo sguardo a chi è rimasto senza diritti e prospettive, soprattutto alle partite IVA, prive di un'adeguata protezione sociale, nonostante rappresentino il motore e il cuore pulsante della nostra economia. Il decreto-legge in esame contempla diverse forme di definizione agevolata dei debiti tributari, soluzioni che contribuiscono a dare corpo alla cosiddetta pace fiscale e che riguardano principalmente le seguenti misure: la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge, che consente ai contribuenti di definire le contestazioni consegnate entro il 24 ottobre 2018, effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata senza sanzioni o interessi; la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui all'articolo 2 del decreto-legge, che consente ai contribuenti di definire gli avvisi di accertamento mediante il pagamento delle sole imposte dovute, senza sanzioni, interessi e somme accessorie; la cancellazione delle cartelle esattoriali per i ruoli sotto i 1.000 euro risalenti al periodo 2000-2010, che consente di cancellare vecchi ruoli di importi molto ridotti che lo Stato non riesce a recuperare da anni e il cui recupero residuo, in ogni caso, porterebbe lo Stato a spendere molto di più di quanto potrebbe guadagnare; la definizione agevolata delle liti pendenti, che prevede che un contribuente vittorioso con l'Agenzia delle entrate in primo grado possa uscire dal contenzioso versando il 40 per cento del valore della lite (chi ha vinto, invece, in secondo grado può versare il 15 per cento del valore della lite); infine, la rottamazione-*ter*, le cui disposizioni sono contenute nell'articolo 3 del decreto. In questa misura si prevede di rottamare le cartelle esattoriali più recenti versando l'imposta originaria con la cancellazione di sanzioni ed interessi. In più, vengono portati da due a cinque gli anni entro i quali saldare le rate dei versamenti. In sede di esame in Commissione abbiamo inoltre esteso la pace fiscale anche a chi ha commesso errori formali. Si potranno, quindi, definire irregolarità in frazioni di obblighi o adempimenti a carattere formale purché non incidano sul calcolo dell'imponibile per imposte dirette, IVA e IRAP. Si dovrà, quindi, pagare una somma di 200 euro per ogni periodo d'imposta cui si riferisce la violazione. La definizione delle irregolarità formali non vale per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Inoltre, con una parte del gettito derivante dalla misura andiamo a rifinanziare il *bonus* bebè, che avrà a disposizione 204 milioni per il 2019 e 240 milioni per il 2020. Costituiamo inoltre un fondo da 474 milioni di euro a valere sul 2019 e 50 milioni a valere sul 2020 per finanziare interventi che riguardano edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico delle aree colpite dalle calamità nei mesi di settembre e ottobre 2018. È stata, inoltre, prevista una serie di misure volte a semplificare e rendere meno impattante l'avvio della fatturazione elettronica tra privati a decorrere dal primo gennaio 2019 con una moratoria delle sanzioni per il primo semestre del 2019. Abbiamo poi previsto l'incompatibilità tra il ruolo di Presidente di Regione e quello di commissario straordinario per il piano di rientro del debito sanitario. In questo modo eliminiamo rischi di commistioni e conflitti d'interesse. Tra i requisiti dei commissari alla sanità da adesso si prevede l'aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture sanitarie pubbliche o private o, comunque, l'aver ricoperto incarichi di particolare complessità anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità. Per quanto riguarda, invece, il lavoro abbiamo previsto altri dodici mesi di mobilità in deroga per i lavoratori delle zone di Termini Imerese e Gela e per tutte quelle zone rientranti nelle cosiddette aree di crisi industriale complessa. inoltre istituito un tavolo operativo per definire una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Questo tavolo sarà composto da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, delle politiche agricole, delle infrastrutture e dell'ispettorato del lavoro, dell'INPS, del Comando dei carabinieri, della Guardia di finanza, delle Regioni e dell'ANCI. Infine, abbiamo approvato un emendamento che getta le basi per la realizzazione di una rete unica delle telecomunicazioni. L'operazione intende favorire lo sviluppo di investimenti in infrastrutture di rete a banda ultralarga ed è funzionale anche alla tutela di valori di rango costituzionale: dalle libertà fondamentali alla garanzia dell'accesso alla rete Internet; dallo sviluppo economico alla coesione sociale e territoriale; dalla crescita digitale del Paese alla tutela dell'occupazione in un settore strategico come quello delle telecomunicazioni. Il tutto, peraltro si inserisce nel quadro dell'agenda digitale che ha l'obiettivo di accelerare la diffusione dell'Internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese. Ha l'obiettivo, entro il 2020, di consentire l'accesso ad Internet a velocità nettamente superiori rispetto a quelle attuali.

della popolazione italiana, oltre che per tutti gli edifici pubblici, poli industriali, aree di interesse economico principali località turistiche e snodi logistici, di perseguire questo obiettivo il decreto apre la strada alla costituzione di una società unica della rete, alla quale verrebbero conferite le attuali reti di Tim e Open Fiber. Oggi l'esistenza di due società comporta la dispersione di risorse che potrebbero essere utilizzate in modo molto più efficiente: una rete unica consente, invece, risparmi consistenti nella definizione delle strategie di investimento nelle reti, senza contare che connessioni più veloci ed efficienti, soprattutto se estese alle attuali zone bianche di mercato - quelle considerate inutili dagli attuali operatori perché troppo poco remunerative rappresentano un risparmio in sé, se si considera la riduzione dei costi che scaturirebbe per l'utenza da una maggiore efficienza della rete. In conclusione, la parte più importante del provvedimento, quella fiscale, contiene norme di definizione agevolata che dovranno rappresentare - unitamente a quelle introdotte per regolamentare i nuovi adempimenti contabili e la semplificazione e razionalizzazione degli stessi una svolta nel rapporto tra Stato e cittadini. In ambito fiscale è necessario superare i luoghi comuni, introducendo una netta distinzione tra l'evasore e colui che, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, non è riuscito, per mera mancanza di liquidità, a versare prontamente le imposte dovute, ampliando, ove possibile, l'utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso di consentire il pagamento in modo dilazionato o con un ritardo sugli stessi pagamenti. Sotto questo aspetto, personalmente non credo sia giusto e corretto definire evasore il contribuente che, pur dichiarando sempre personalmente non credo sia giusto e corretto definire evasore il contribuente che, pur dichiarando sempre e da sempre il proprio reddito, conformemente all'ordinamento fiscale vigente, in un contesto di assoluta legalità è stato costretto, da problemi legati alla liquidità, a rinviare o omettere il versamento delle imposte. Spesso si è ritenuto di gran lunga più agevole cavalcare la facile indignazione sull'argomento evasione, legata soprattutto alla lettura della realtà offerta da soggetti che possono contare su redditi che consentono una maggiore sicurezza economica; sicurezza che i lavoratori autonomi, i professionisti e le imprese hanno visto invece vanificata negli ultimi anni. Concludo, ringraziando la Commissione: i funzionari della Commissione, il presidente Bagnai, i rappresentanti dal Governo e i colleghi commissari di tutte le parti politiche che hanno partecipato attivamente alla discussione del decreto-legge attraverso un lavoro puntuale, con l'obiettivo comune di migliorare il provvedimento. Queste misure in ambito fiscale rappresentano un primo passo: sono misure necessarie anche per indicare la direzione che vogliamo seguire: la tutela della dignità dei contribuenti, dei lavoratori, delle imprese, la dignità di coloro che da sempre hanno creato la ricchezza nel nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi M5S

presto la mia voce allo spirito civico e impegnato che si sta risvegliando nel nostro Paese per dire che siamo preoccupati. Parlo del decreto-legge fiscale facendo un passo indietro

punti base; i BTP hanno perso l'11 per cento del loro valore, gli investitori, i *retail*, stanno fuggendo dalla sottoscrizione del nostro debito pubblico, e infatti l'asta che è andata deserta la scorsa settimana,

di questo Esecutivo di vedersi cristallizzato in un'altra asta deserta. La Banca d'Italia ha certificato che la ricchezza degli italiani è diminuita del 3,5 per cento in questa prima parte della XVIII legislatura

noi invece diciamo che è successo qualcosa di peggio, perché tutto questo collasso è avvenuto solo a chiacchiere, perché i cosiddetti numerini devono ancora essere approvati: la legge di bilancio deve ancora essere approvata

perché impiega 37 miliardi per porre in essere misure assistenziali, per mantenere l'IVA così come è, per non abbassare le tasse e per mortificare ancora una volta il pubblico impiego, stanziando solo un miliardo per rinforzare le Forze dell'ordine, gli addetti alla giustizia. Le tasse non vengono diminuite, se non per l'1,2 per cento di fortunate partite IVA che pagheranno molto meno di coloro che invece nel lavoro pubblico avranno redditi uguali.

dalla mini Ires, avrà un saldo negativo sui contribuenti, sulle imprese, sull'asse portante del nostro Paese. Inoltre, si

è prevista qualche sanatoria, qualche rottamazione, qualche condono. Oggi stiamo parlando di questo perché il decreto fiscale si compone di tre parti:

per emendamento, bypassando tutto il dibattito parlamentare, le audizioni e l'unica cosa seria che c'è in questo Parlamento, cioè la riflessione approfondita sulle cose importanti da fare per il futuro di questo Paese.

pressoché senza fare gettito. Si è persa veramente una grandissima occasione, perché un vero decreto-legge fiscale avrebbe dovuto affrontare ciò che è stato detto essere urgente, cioè una vera riforma del fisco. Per noi una vera riforma del fisco è questo: introdurre una revisione profonda delle *tax expenditure*; introdurre una prima fase della *flat tax*, che non fa arrabbiare nessuno introducendo una *no tax area* per mantenere la progressività dell'imposta e diminuendo le due aliquote più basse in modo da aiutare subito, urgentemente, le classi sociali più in difficoltà in questo momento. È stato fatto tutto questo? No, naturalmente;

principalmente in cinque modi. Abbiamo fatto notare che è stata data la possibilità di condonare i processi verbali di constatazione, gli avvisi di accertamento, le liti pendenti: è stata quindi data la possibilità di condonare a coloro che non avevano versato. L'unica cosa che non è stato possibile fare è stato dare la possibilità a quelli che avevano regolarmente versato, e che hanno commesso degli errori formali o non hanno potuto versare le imposte per difficoltà, cioè i beneficiari - diciamo così - di avvisi bonari, di condonare. Questo non è stato possibile farlo. Non è stato possibile nemmeno uniformare uniformare il trattamento di chi aderiva alla rottamazione-*ter*. Si sono fatte delle finestre *random*, temporali, che differenziano contribuenti che sono nelle stesse identiche situazioni. quindi coerenza. Poi ci si era dimenticati completamente del settore pubblico, delle imposte degli enti pubblici, della Tari, dell'IMU. Abbiamo suggerito un emendamento, che è stato recepito dal Governo. Sulle liti fiscali si era persa la bussola del realismo, perché è realistico pensare che il contribuente sia parzialmente vittorioso in una contesa con il fisco? Noi abbiamo dato la possibilità di definire anche queste posizioni. Poi abbiamo dato la possibilità di definire l'unica cosa che si doveva fare, cioè le violazioni alle dichiarazioni che non incidevano sui tributi, cioè di coloro che hanno versato tutto, ma che hanno commesso degli errori meramente formali. Questo ora è possibile farlo. Abbiamo lottato - questo devo dirlo - invano, drammaticamente, per evitare l'allungamento dei termini di accertamento. Perché un condono che è stato presentato come nobile strumento di pacificazione fiscale deve provocare *erga omnes* un allungamento dei termini di accertamento? Questo è inaccettabile nel ristabilire un equo rapporto tra fisco e contribuente.

umanamente sostenuti in questa battaglia, nell'interesse - almeno da parte nostra - dei contribuenti, per evitare che questa visione in cui il contribuente è solo un evasore passasse del tutto. Noi non siamo d'accordo su questa visione. Ciò su cui ci siamo assolutamente trovati d'accordo è la fatturazione elettronica. La fatturazione elettronica non può essere un archetipo di uno strumento per fare cassa su chi produce. l'idea *sui generis* che questo Governo ha del mondo produttivo, che gli nega l'importanza e la dignità di essere veramente la spina dorsale di questo Paese. Una fatturazione elettronica che non ha aiutato che non ha aiutato eliminando le sanzioni per tutto il 2019, che non ha spostato il termine di introduzione della fatturazione elettronica per i soggetti più piccoli, che non ha nemmeno agevolato l'acquisto di strumentazione *software* e che non ha agevolato la formazione del personale. Come può uno Stato pretendere di introdurre un obbligo a carico dei contribuenti quando esso stesso

ringrazio lei e l'Assemblea per l'attenzione che viene riservata a questo argomento, che non è un argomento qualsiasi. È l'argomento in ragione del quale il nostro sistema-Paese provvede al potenziamento delle risorse finanziarie almeno dovrebbe essere questa la rubrica della norma. La denominazione del decreto-legge ci fa pensare che questo strumento dovrebbe essere quello che consente al sistema-Paese di avere certezza fiscale, funzionalità tributaria e provvista di gettito, per far sì che le decisioni, i diritti, le opportunità e le comodità trovino - come mi piace dire - copertura. si configura in Italia il sistema tributario, in questo momento, cioè prima della vigenza del decreto-legge di cui ci occuperemo, spero con crescente attenzione:

pagano le tasse, pari al 76 per cento della platea degli italiani che hanno dovere e diritto; 840 miliardi sono la raccolta tributaria e contributiva. Nel 2017 le azioni del nostro sistema-Paese hanno portato a un recupero di evasione fiscale pari a 20 miliardi di euro.

Abbiamo anche determinato una riduzione della pressione fiscale pari a - 1,1 per cento. Qual è il problema aggiuntivo da fronteggiare con lo strumento denominato in passato decreto-legge Fare in modo che continui la lotta all'evasione, poiché c'è ancora un margine di lavoro possibile pari a 120 miliardi di euro. Abbiamo fatto le audizioni, cari colleghi, non per abbellire il tempo del non lavoro in Commissione, ma perché sono servite per aumentare elementi, capacità conoscitiva e robustezza delle nostre decisioni: Corte dei conti, nella figura del Presidente (non il centro studi privato, ma il presidente della Corte dei conti Buscema); l'Agenzia delle entrate a livello nazionale, quella che avete rinnovato; la Guardia di finanza, nella figura del vertice e poi il capo dipartimento del MEF fiscalità. Tutte e quattro queste figure ci hanno detto che la fatturazione elettronica è un'infrastruttura che concorre alla riuscita del nostro sistema tributario. Noi, nei 26 articoli del decreto-legge denominato decreto-legge fiscale, abbiamo trovato tutto salvo che la scommessa per far funzionare di più la fatturazione elettronica. Abbiamo annacquamenti e tentativi di sviare la capacità di insediamento e potenziamento della fatturazione elettronica. Questo

specie di paniere, di contenitore che deve soddisfare segmenti di portatori di interessi egoistici. Cito un caso che mi aiuta molto e, se fossi in un tribunale, vincerei la causa: quanto si è fatto sulle sigarette elettroniche. della giustizia costituzionale, che dice che quella tassazione è giusta, che va esatta, pretesa, introitata e messa nel circuito degli investimenti, il legislatore organizza uno sconto, una donazione, un'amicalità eccessiva; altro che *compliance*! Amicalità, gelatinosità che toglie 187 milioni di euro.

La donazione che si è fatta sulle sigarette elettroniche, a mio avviso, è bene che diventi oggetto di un convegno, di un dottorato, di un corso di laurea per capire come non si fa il decreto-legge fiscale, come non si costruisce la regola fiscale nei confronti di chi deve e ha obbligatorietà tributaria. Ma occorre parlare anche dell'articolo 9,

professore di diritto pubblico Giuseppe Marazzita, figlio dell'avvocato Nino Marazzita che si batte per i cittadini consumatori, in un corso di laurea dedicato al diritto pubblico, sostiene che è un'originalità propria di questa stagione deliberativa, ministeriale, politica, un decreto-legge che vede due volte la luce. Perché vi è stata una doppia deliberazione? Qual era il tema che faceva la differenza tra prima e seconda stesura? L'articolo 9, quello della istanza dichiarazione integrativa speciale, che consentiva un condono indigeribile anche a vigenza del contratto di Governo. Governo. Quel condono di cui all'articolo 9, infatti, era il grimaldello che ha crepato il contratto di Governo, perché nei fatti poi è stato tolto, tolto, cancellato, rimpicciolito, immiserito, reso compatibile con la veduta di tutta la coalizione. Ma qual era l'originalità di quell'articolo 9, che non c'è più, ma che noi dobbiamo tenere a mente, come una stigmate di ciò che non si deve fare più? Si determinava la *flat tax* per l'evasore. La *flat tax*, che è un grande capitolo del contratto di Governo, di questa riuscita di cui siete stati capaci sul piano elettorale, solo per gli evasori, compare in ragione della manina e scompare perché scompare la manina; la *flat tax*, con l'aliquota al 20 per cento solo per questi fortunati. Ma perché? Qual è la visione del rapporto tra cittadini e Stato, tra contribuente e diritto-dovere, obbligatorietà? È su questo che abbiamo lavorato in Commissione. In Commissione non siamo stati elementi di arredamento o di conflitto: abbiamo cercato, uno per uno, di cucire le gambe a un diritto tributario che non può essere invalidato.

che il perfezionamento contrattuale tra contribuente e ordinamento tributario non si può realizzare con il pagamento della prima rata. La prima rata, che perfeziona il contratto tra contribuente e ordinamento tributario, fa saltare tutto il seguito degli adempimenti. Non a caso la rottamazione*-bis* ha conosciuto una sorta di liquefazione, perché le parole «da luglio a seguire» hanno fatto capire che ci sarebbe stata una rottamazione-*ter*.

Franco Gallo dice che non si può scherzare col diritto tributario; le parole fanno male, disorientano e in qualche modo destabilizzano. Cosa si è creato a luglio? Circolando la voce che ci sarebbe stata la sanatoria, il giubileo fiscale, la gente ha smesso di pagare sono mancate le entrate. Se mancano le entrate, il sistema Paese non ce la fa ad essere Paese, Stato e Nazione. Altro che convegni sulla sovranità, sul nazionalismo e sul di più che deve fare il sistema Paese. Mettiamoci d'accordo allora; il decreto-legge fiscale provvede alla provvista e poi la legge di bilancio alloca. Questo provvedimento è una specie di arca dove c'è tutto: autostrade, autorità portuali,

Signor Presidente, abbiamo scelto di presentare la questione pregiudiziale di costituzionalità perché non possiamo rassegnarci al fatto che ormai

nostro esame. Non vogliamo rassegnarci perché non è assolutamente possibile continuare ad accettare quasi supinamente una

da parte di costituzionalisti ogniqualvolta qualche maggioranza di Governo presenti una bozza di riforma costituzionale, ma poi tutto continua nello stesso modo.

l'articolo 77 della Costituzione, alcuni provvedimenti, per esempio, non entrano in vigore subito, ma sono spostati in là nel tempo. Pensiamo ad esempio

stata indicata con chiarezza anche dallo stesso Comitato per la legislazione della Camera. Accade sempre più frequentemente che il Consiglio dei ministri approvi, come si dice in gergo, la camicia

cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Quella norma, nello specifico, intanto intanto introduce una forma di disparità, tale per cui chi ha chiuso la rottamazione prima, magari accettando soltanto le due rate, oggi è escluso; un'altra platea di contribuenti, invece, che magari non ha ancora concluso la fase della rottamazione

un'altra. E secondo voi, questo è il rispetto dell'articolo 53 della Costituzione, delle persone perbene e della maggior parte dei contribuenti, che sono quelli a cui il prelievo viene fatto direttamente? Io credo assolutamente di no. Per tutti questi motivi, caro Presidente

vogliamo sottoporre alla trattazione del Parlamento la questione pregiudiziale che sentiamo di proporre relativamente al decreto-legge n. 119 del 2018. Premesso che vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame, per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso del decreto legge,

trasformando il decreto-legge in un insieme di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale e prive di uno scopo unitario. Il fatto, poi, che le misure previste dal decreto-legge siano tra loro estremamente eterogenee costituisce di per sé l'evidente dimostrazione della carenza del requisito della straordinarietà del caso e della necessità e dell'urgenza di provvedere. Infatti, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, i presupposti per l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. Come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012, «ove le discipline estranee alla *ratio* unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risultano invece in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei». consideri che tale ultimo caso riguarda con tutta evidenza il presente decreto-legge, che palesa una manifesta eterogeneità delle materie disciplinate: vi sono infatti le numerose misure di condono e sanatoria, vi è tutta una serie di misure riguardanti le Ferrovie dello Stato, la cassa integrazione per riorganizzazione o crisi aziendale e l'incremento del fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali previsto nella legge quadro n. 145 del 2016, il cui finanziamento ordinario certo non può essere considerato un caso straordinario di impellente necessità e urgenza. La puntuale giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171 del 2007 e 128 del 2008...

della Carta fondamentale non può evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta». In tali pronunce la Consulta ha peraltro sottolineato che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva, ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte. Si consideri che le recenti polemiche sorte in seno all'Esecutivo sull'inserimento di norme di condono fiscale nel decreto-legge, che non sarebbero state esaminate e approvate dal Consiglio dei ministri, è una diretta conseguenza di una modalità di legiferare basata sull'abuso dei decreti-legge. Pertanto, se si vogliono evitare questi inconvenienti che minano la credibilità dell'Esecutivo, le forze di maggioranza dovrebbero limitare il ricorso alla decretazione di urgenza, come purtroppo avvenuto spesso in questa legislatura, e presentare le loro proposte in disegni di legge ordinari, come prescrive la Costituzione, assumendosene la piena responsabilità politica. Le Camere le discuteranno e le approveranno, con la pubblicità che caratterizza i lavori parlamentari a garanzia della trasparenza, della collegialità e della democraticità dell'*iter* legislativo ordinario, che la Costituzione assegna al Parlamento quale organo rappresentativo di tutti i cittadini. del fatto che anche sul merito stesso del provvedimento emergono forti perplessità: la prima riguarda la più complessiva tenuta del sistema tributario, che il decreto-legge in esame mette di fatto in discussione. Si tratta di un articolato pieno di sanatorie e condoni, che minano la credibilità dell'intero sistema tributario di fronte ai cittadini e che rischiano di minare gravemente le future entrate fiscali. La seconda grave ferita al nostro sistema fiscale è costituita dalla caratteristica di queste misure definitorie, come ad esempio quella prevista dall'articolo 8 del decreto-legge in materia di definizione agevolata delle imposte di consumo. L'articolo 8 contiene la definizione agevolata dei debiti tributari maturati a titolo d'imposta sui consumi con il versamento del 5 per cento Si tratta in realtà di una sanatoria fiscale con un maxisconto, prevista per gli operatori del settore della produzione e commercializzazione della sigaretta elettronica: un trattamento diverso e quindi una evidente e manifesta violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, una discriminazione palesemente irragionevole, perché penalizza i contribuenti che adempiono alle loro obbligazioni tributarie e che pagano per intero l'imposta e premia in modo del tutto ingiustificato chi non ha dichiarato e pagato per tempo quanto dovuto. Una tale irresponsabile violazione del principio di uguaglianza e smentita del principio di progressività del sistema tributario discrimina i contribuenti onesti e rischia di spingere tutti i cittadini defraudati da una tale ingiustizia a violare in futuro le norme tributarie e a non pagare le imposte dovute in ragione di sanatorie che premiano i comportamenti illeciti. L'intervento previsto all'articolo 3 si configura come un palese danno a carico del bilancio pubblico. In sostanza, le nuove norme sulla definizione agevolata (rottamazione-*ter*) dei carichi affidati all'agente di riscossione ripropongono norme già vigenti, che, in ragione delle varianti di maggiore favore in termini di rateizzazione e di riduzione degli interessi (che si pagheranno allo 0,3 anziché al precedente 2 cento) e delle sanzioni, hanno l'effetto di produrre minori entrate all'erario sulla riscossione ordinaria e sulla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione attualmente in corso. Concludo con una riflessione sull'articolo 4 relativo allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati

per gli enti territoriali coinvolti. Al riguardo sarebbe stato più rispettoso dell'autonomia locale, concedere, in luogo dello stralcio, un termine all'ente creditore per la riattivazione del credito non prescritto mediante la notifica di un'ingiunzione di pagamento entro una data prestabilita, salvaguardando per i bilanci degli enti locali coinvolti. Per tutte le motivazioni che abbiamo elencato e le valutazioni fatte, chiediamo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 886.

al potere legislativo attribuito al Parlamento. Abbiamo poi una eterogeneità di misure che ne caratterizzano il contenuto. il contenuto. Sono state più volte richiamate sentenze della Corte costituzionale che hanno ben illustrato, hanno ben indicato la strada che dovrebbe essere seguita dal Governo per poter utilizzare questo strumento

che tenta di mettere in sicurezza una serie di benefici, o addirittura di ampliare alcuni benefici per categorie limitate, senza che vi sia una connessione chiara ed evidente fra le differenti misure. È uno spezzatino. Sono misure che, peraltro, portano anche a discriminare

quei contribuenti che adempiono alla loro obbligazioni tributarie, che pagano per intero l'imposta e premia invece in modo ingiustificato chi non ha dichiarato e pagato chi non ha dichiarato e pagato per tempo quanto dovuto; questo è grave che avvenga da parte dello Stato. Come è stato illustrato nella relazione di minoranza, il fatto che questo decreto-legge abbia visto la luce due volte due volte evidenzia come il Governo stesso abbia avuto serie difficoltà nell'elaborare la propria strategia ma di fatto la strategia non c'è. La ragione per cui è stato riapprovato dal Consiglio dei ministri è perché all'interno della maggioranza si era creato un evidente *vulnus*

quali siano le ragioni e se sussistano le motivazioni che portano oggi a votare un decreto-legge che non aveva ragioni di effettiva urgenza perché la trattazione delle misure che contiene poteva essere oggetto di un ordinario disegno di legge. Addirittura alcune di queste misure potevano tranquillamente essere inserite nella legge di bilancio che l'altro ramo del Parlamento ha iniziato a discutere. Crediamo Crediamo che il rispetto che si deve alla Costituzione e alle modalità con le quali il Governo è chiamato ad intervenire nella funzione legislativa debbano far ragionare tutti in quest'Aula sul fatto che ragioni per proseguire nell'esame del decreto-legge. Se entriamo poi nel merito, come è stato evidenziato nelle relazioni e nelle questioni pregiudiziali, abbiamo una serie di elementi critici, da un lato discriminatori - come è stato richiamato - ma dall'altro anche

troppe materie, tra loro diversificate, senza che emerga in maniera chiara dove sia l'urgenza di dover procedere con un decreto-legge, anziché con provvedimenti legislativi ordinari

condannato, che è quello di essere furbi in relazione alle proprie responsabilità fiscali nei confronti dello Stato, comprendiamo che questo è un decreto-legge che, anche dal punto di vista della pedagogia politica, dovrebbe essere subito accantonato e non dovrebbe essere discusso.

di recupero dell'evasione fiscale: sono state già citate e non è la prima volta che ciò emerge. Quando abbiamo approvato il rendiconto del 2017 è stato certificato, da parte del Governo, che l'evasione fiscale recuperata aveva assunto dimensioni considerevoli. Questa è l'azione che dovrebbe essere incentivata da parte del Governo e che dovrebbe essere ulteriormente sviluppata, ma di questa misura non vi è traccia. L'altra misura è quella che dovrebbe andare in maniera strutturata a proseguire nella riduzione della pressione fiscale e invece, nuovamente, il decreto-legge in esame non fa che piccoli ritocchi - come è stato fatto notare nella discussione misure che vanno a dare piccoli benefici a porzioni limitate di contribuenti. Nulla a che vedere con le azioni intraprese dai Governi precedenti e che hanno consentito

A mio avviso è il contrario, proprio per il fatto che il decreto-legge non va a tutelare la dignità dei lavoratori che pagano ordinariamente le tasse, non va a tutelare la dignità dei contribuenti che regolarmente adempiono ai propri doveri doveri fiscali, non va a tutelare la dignità delle imprese che ordinariamente e con fatica pagano le tasse. Queste considerazioni ci fanno dunque dire che il decreto-legge in esame non è per la dignità e la correttezza del rapporto tra contribuente e Stato. Per queste ragioni crediamo che non vi siano motivazioni per procedere nell'esame di questo decreto-legge e il nostro invito al Governo è di ritirarlo e di procedere lavorando in Parlamento con provvedimenti che indichino davvero l'indirizzo dell'Esecutivo e del Paese. Indirizzo che deve essere quello di un recupero dell'evasione costante, di un rapporto tra lo Stato e i contribuenti che sia corretto, orientato in maniera costante

non un condono, come è stato detto, ma un nuovo rapporto col fisco, basato su reciproca fiducia. In esso è inserita la rottamazione-*ter*, a condizioni decisamente più favorevoli rispetto a quella precedente; un arco temporale più ampio; tassi di interesse ridotti; lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: debiti ovviamente tributari, che riguardano le cartelle dal 2000 al 2010; una definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la regolarizzazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche attraverso agevolazioni: un settore, quello dello sport, che è in grande difficoltà e che, a nostro giudizio, anche a livello politico va sostenuto. Se non lo sosteniamo, infatti, poi andate voi a dire ai nostri ragazzi che

questione dell'IVA, dove il concessionario committente può detrarre l'imposta nella liquidazione relativa al mese in cui la fattura è stata emessa. Anche questa è una richiesta più volte sollecitata dai nostri imprenditori e dai nostri artigiani. il sostegno alle agevolazioni per il sistema dell'autotrasporto, che è in difficoltà, con un finanziamento legato anche al sistema portuale. Vi è il famoso articolo 9, la reintroduzione del *bonus* bebè, addirittura con delle agevolazioni, perché c'è il 20 per cento in più rispetto al secondo figlio. Quanto alle agevolazioni sulle sigarette elettroniche, perché si devono pagare più tasse se alla fine fanno meno male? Questo fatto qualcuno qui dentro, prima o poi, me lo dovrà spiegare. condono, ma è una regolarizzazione degli errori formali. Vogliamo andare a dire ai nostri cittadini che, per errori formali nella compilazione della dichiarazione dei redditi, devono pagare sanzioni? *(Applausi

Vogliamo dimenticare il sostegno alle popolazioni che sono state colpite dalle ultime devastazioni? Anche qui, c'è un contributo non da poco. Abbiamo fatto diversi interventi, richiamando certamente un intervento del Governo stesso per aiutare e sostenere queste popolazioni; e abbiamo visto che le devastazioni sono state tante. Per chiudere, ricordo il tema della banda

a presentare la posizione di Fratelli d'Italia. Abbiamo ascoltato le motivazioni contenute nelle pregiudiziali presentate ai sensi dell'articolo 93 del nostro Regolamento ma, seppur potremmo

ribadendo quanto già sostenuto in Commissione per quanto è condivisibile (molto poco) e per quanto non è condivisibile (la gran parte, se non la totalità). Fratelli d'Italia ribadisce, con il suo voto di astensione alle pregiudiziali presentate, una sua opposizione patriottica, fatta sempre nell'interesse e nel bene del Paese prima di tutto.

a un decreto-legge fiscale che oggi possiamo davvero rinominare decreto *omnibus*, ma per niente fiscale; dopo diverse giornate, nelle quali Fratelli d'Italia ha cercato, con la serietà che vuole contraddistinguerci, di portare un contributo senza fare mai ostruzionismo. Ci vantiamo di non aver sprecato un minuto del nostro tempo nell'ostruzionismo, ma di aver cercato, con forza, con impegno, con determinazione, di migliorare il decreto-legge Un provvedimento che, come avrò modo di dire più tardi quando farò un'analisi in sede di dichiarazione di voto, non ci soddisfa. Vorrei, però, in questo contesto di discussione generale soffermarmi su un tema che certamente non è fiscale, visto che, come detto, quello che esaminiamo oggi è un decreto *omnibus*, ma che avrebbe potuto almeno dare le «stellette» a questo decreto-legge.

con una vera voglia di ridare fiato al credito nazionale, quel credito nazionale che - lo ripeto - è ormai sparito dalla nostra Patria e oggi è controllato, come un cavallo di Troia, dalla finanza internazionale.

il credito cooperativo, quelle casse rurali che noi tutti, nelle nostre periferie, nelle nostre vallate, abbiamo sempre visto come una risorsa come una risorsa della mutualità, nella territorialità, nella capacità di rispondere davvero ai problemi e alle esigenze degli artigiani, dei contadini e delle piccole imprese.

Fratelli d'Italia si è impegnata cercando di proporre degli emendamenti e cercando di fare proprie anche le posizioni della Lega, che inizialmente erano volte a dare un segnale di discontinuità;

scalata della *holding* delle casse rurali, quindi oserei dire che purtroppo ho la certezza che nei prossimi due o tre anni il nostro credito cooperativo non sarà più patrimonio della nostra Nazione.

interverrà la capogruppo, con la logica di una società per azioni, magari controllata anche da strumenti finanziari stranieri. In sostanza, il cavallo di Troia rappresentato dal sistema bancario,

italiana. Voglio concludere questo mio intervento ricordando peraltro che ci sono dei gravi profili di incostituzionalità che sono stati ignorati, e voglio quindi sperare che i prossimi mesi possano comunque portare a questo Parlamento la volontà di porre rimedio in qualche modo a questo disastro che coinvolge il credito nazionale; lo chiedo, prima ancora che da senatore, da esponente politico, da professionista, da cittadino, da socio delle casse rurali.

Signor Presidente, colleghi senatori e colleghe senatrici, il provvedimento che siamo oggi chiamati a votare rappresenta un passaggio preliminare e importante per la prossima legge di bilancio. Siamo di fronte, e abbiamo il dovere di gestire, uno spropositato numero di ruoli iscritti e non incassati, che rappresentano un enorme fardello per lo stato patrimoniale e per gli equilibri finanziari della Nazione. Un fardello che affligge l'Italia ormai da decenni e che ha contribuito non poco a ingenerare la grave situazione finanziaria cui oggi siamo chiamati, con non poche difficoltà, a fare fronte, visto che finora i risultati degli interventi legislativi precedenti si sono dimostrati del tutto inadeguati. infatti noto come le mancate riscossioni pesino sul bilancio dello Stato e come tali pesi influenzino in maniera determinante le scelte del Parlamento e le politiche legislative che esso si propone di perseguire. Tra le mancate entrate del bilancio dello Stato, infatti, oltre ai ruoli iscritti e non incassati, si deve considerare anche l'enorme valore rappresentato dal sommerso economico che, secondo l'ultimo rapporto ISTAT, ammonta a circa 210 miliardi di euro, cioè più o meno il 13 per cento del nostro PIL. Parliamo, poi, di una evasione fiscale che, stando ai dati fomiti dal MEF lo scorso ottobre, ci costa circa 110 miliardi di euro. A ciò si aggiungono gli sconcertanti dati dell'ultimo rendiconto di gestione, appena approvato, che, come sottolineato anche dalla Corte dei conti, evidenziano residui attivi per un valore di circa 204 miliardi dì euro; dato, questo, che mette ancora di più in risalto, come se ce ne fosse bisogno, le criticità a cui accennavo prima e che diventa ancora più drammatico se si considera che al netto delle presunzioni e apprezzamenti prudenziali esso ammonta a circa 900 miliardi di euro, soltanto per la

dati confermano la perdurante difficoltà dello Stato a stabilire un rapporto positivo con i contribuenti, un rapporto che si riveli in grado di invogliare e facilitare quest'ultimi a versare le imposte dovute, anziché alimentare una crescente conflittualità su un tema di vitale importanza per la sopravvivenza stessa del Paese (parliamo dell'equilibrio finanziario dello Stato). Sono dati che ad oggi fanno tremare le vene ai polsi e da cui dobbiamo ripartire, consapevolmente, per adottare tutte quelle misure legislative che sono indispensabili, e sempre più urgenti, per migliorare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale patrimoniale dello Stato, così da renderlo immune rispetto a qualsivoglia speculazione finanziaria. È solo così che si potrà liberare l'Italia e gli italiani dallo spauracchio dello *spread*. Lo *spread* spaventare soltanto uno Stato che ha una situazione finanziaria precaria: è questo il vero problema dell'Italia, al quale dobbiamo porre rimedio nel più breve tempo possibile. Ed è proprio in questa direzione che muove il provvedimento oggi al nostro esame: chiudere con un ammasso di situazioni debitorie che sono state portate avanti per decenni dallo Stato come una sempre più insostenibile zavorra, per poi continuare questo percorso che avrà come obiettivo prioritario quello di migliorare il rapporto tra il cittadino-contribuente e lo Stato. Si tratta di una vera e propria riappacificazione, graduale e continua, che passa attraverso provvedimenti legislativi tesi a rivedere le logiche del fisco in un'ottica sempre meno vessatoria e, contemporaneamente, il funzionamento stesso della pubblica amministrazione, soprattutto in una prospettiva di miglioramento della *performance*. A tale proposito, aggiungo che nelle prossime giornate discuteremo in Aula il disegno di legge concretezza. Pertanto dobbiamo scrivere un nuovo capitolo che ridisegni il rapporto tra fisco e contribuente, per aiutare quest'ultimo che ancora oggi è costretto a fronteggiare da solo un sistema tributario denso di insidie, adempimenti, scadenze sempre più frequenti e ravvicinate, nonché vere e proprie ritorsioni. Infatti, negli ultimi decenni chi è stato chiamato alla guida del Paese ha fatto poco o nulla per migliorare l'efficacia e l'efficienza del funzionamento dello Stato, generando un *trend* finanziario negativo confermato purtroppo dallo stato patrimoniale del bilancio, che per i dati finanziari è impietoso, con carattere tendenziale negativo - che vede nel crescente debito pubblico la sua più grande e inconfutabile prova. Il debito pubblico è infatti il vero peccato capitale che viene scaricato sui cittadini attraverso un sistema tributario sempre più aggressivo e colpevolizzante. Con la conversione di questo decreto-legge fiscale abbiamo la possibilità di iniziare un percorso in cui i contribuenti possano uscire da questo stato di paura e, soprattutto, muovere un primo passo verso un ripensamento della fiscalità che, finalmente, riconosca nel cittadino un contribuente e non più un imputato da rincorrere e vessare, ridando forza e vitalità a un rapporto Stato-cittadino oggi sin troppo deteriorato. Con la conversione di questo decreto-legge fiscale compiamo soprattutto quel primo passo necessario per una riappacificazione tra Stato e cittadino, a cui però non bisogna guardare come fosse isolato o il frutto di un mero provvedimento estemporaneo. È questo, infatti, un passo che deve essere letto insieme al ripensamento del funzionamento della pubblica amministrazione; un ripensamento che possa portare lo Stato nelle condizioni di garantire una maggiore efficacia ed efficienza ed efficienza nella fornitura di quei servizi che sono degni delle migliori società civili e che lo Stato è chiamato ad assicurare a tutti i cittadini. Questo è l'impegno che il MoVimento 5 Stelle ha preso verso l'Italia e verso i cittadini italiani.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è il primo provvedimento di attuazione della Nota di aggiornamento del DEF, il cui contenuto è fondamentalmente costituito dalla materia fiscale. In particolare, rappresenta il primo passo per ristabilire un rapporto di fiducia tra fisco e contribuente. Le numerose norme che abbracciano un'ampia gamma di ricomposizione di liti, anche solo potenziali, sono destinate ad avere effetti positivi sul decongestionamento degli organi di giustizia tributaria, nonché degli uffici finanziari presso i quali ingenti risorse umane - e conseguentemente finanziarie - vengono distolte dagli impegni relativi alla gestione del contenzioso per essere rivolte ad altre attività più proficue. Quanto alla platea dei contribuenti, gli stessi si troveranno liberati dal peso, a volte insostenibile, derivante da imposte, tasse, interessi e sanzioni iscritte in ruoli di vecchia data, ma ancora costituenti concreti impedimenti all'esercizio delle attività economiche alla luce del sole, come nel caso del piccolo commerciante o del piccolo artigiano, schiacciati dalla crisi e impossibilitati a onorare vecchi debiti fiscali, se non mettendo a rischio di chiusura la propria modesta attività. Dal lato della fatturazione elettronica ci si è attivati al fine di porre rimedio alle criticità nell'ambito della tutela della *privacy*, rinviandone l'obbligo di emissione per gli operatori economici che trattano notoriamente dati sensibili, come i professionisti del settore sanitario, già peraltro peraltro obbligati alla trasmissione dei dati all'interno del sistema tessera sanitaria. Tale proroga non incide quindi sulle previsioni di entrata formulate già dal passato Governo, permettendo di recepire le osservazioni del Garante in tempi adeguati. Peraltro, si evidenzia come l'obbligo della fatturazione elettronica riguarderà alla fine, nel 2019, una platea per quanto possibile limitata di contribuenti, tenuto conto dell'esclusione degli operatori economici sanitari, dei forfettari soggetti a *flat tax*, degli esercenti al minuto, soggetti allo scontrino fiscale, nonché degli altri regimi speciali, quali quello vigente nel settore agricolo. Siamo consapevoli delle problematiche che comporterà la fatturazione elettronica, ma non dimentichiamo che l'obbligo della fatturazione elettronica è un'eredità lasciataci dal precedente Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. infatti è stato imposto come termine iniziale il 2019, prevedendo maggiori entrate per ben 2 miliardi di euro, quale conseguenza dell'emersione del nero. Ed è tale previsione di maggiori entrate che ha, di fatto, impedito la possibilità di una proroga, pena una variazione negativa delle entrate, non colmabile nel breve periodo con il reperimento di altre diverse risorse. Si è ulteriormente agito con norme di semplificazione degli adempimenti fiscali incombenti sui contribuenti, sulla scia di quanto già intrapreso col decreto-legge dignità; il tutto teso a ridurre i costi delle imprese. Si è agito per venire incontro all'esigenza dei contribuenti al fine di mitigare l'impatto della novità, con consistenti riduzioni delle sanzioni relative a violazioni che non comportino evasione d'imposta, prevedendo maggiori tempi per l'emissione delle fatture e semplificazioni in tema di annotazione delle stesse. Anche nel comparto della giustizia tributaria digitale si è prevista una razionalizzazione delle procedure, con l'introduzione a regime delle modalità telematiche. Si è ritenuto di dover intervenire anche nel senso di un contenimento dell'imposizione fiscale gravante sulle cosiddette sigarette elettroniche, al fine di superare il complicato calcolo di equiparazione della sigaretta tradizionale con quella elettronica, che ha provocato l'esodo delle aziende produttrici di dispositivi e di liquidi all'estero. Con lo sgravio, inoltre, si va in una direzione di incentivazione all'abbandono della sigaretta tradizionale. Al collega D'Alfonso, relatore di minoranza, faccio notare che, sì, si è messo mano a tante, diverse questioni, contraddizioni e situazioni frutto dell'operato di precedenti Governi. E non tutto è stato ancora risolto, ne siamo consapevoli: non basta ancora. Abbiamo iniziato ad arginare le conseguenze di politiche congeniate contro la classe imprenditoriale e contro il contribuente. Concludendo, il provvedimento va davvero nel senso della pace fiscale: contribuenti che non hanno pagato le tasse perché oggettivamente impossibilitati, contribuenti che hanno dichiarato e sono rimasti imbrigliati nelle maglie del fisco. Ebbene, colleghi, non abbiamo ancora raggiunto i sei mesi di Governo, eppure siamo qui a votare un provvedimento in piena linea con quanto promesso. Questo Governo sta lavorando per onorare quanto promesso, passando cosa rara in politica - dalle parole ai fatti.

nel Consiglio dei ministri, che lo ha varato per due volte, poi in Commissione, un decreto-legge *omnibus*, in cui vi è tutto e il contrario di tutto. Vi sono norme di grande rilevanza, almeno nella prospettiva che indicano, come la società unica della rete, che viene introdotta come concetto con un emendamento surrettizio in un provvedimento che si chiama decreto fiscale. Cosa c'entri la rete con il decreto fiscale

ovviamente è un fattore strategico anche per quanto riguarda gli assetti industriali del Paese, e con altre questioni, come quella del *bonus* bebè, di cui vi eravate dimenticati nella manovra. È un decreto-legge *omnibus*, non è più un decreto fiscale. Peraltro lo stesso relatore, nel suo intervento,

è contestata in sede europea. Avete venti giorni per cambiare la legge di bilancio e la state cambiando. Con quale obiettivo? Da quello che si legge, l'unico obiettivo che vi interessa

dell'infrazione. Sembra un Governo di ripetenti, ripetenti nella vita, ripetenti nel Governo. Chiedete il rinvio a settembre dell'infrazione e attraverso che cosa?

Se cambiate la manovra nella sostanza, se, per esempio, il reddito di cittadinanza diventa una risorsa data all'impresa per assumere anche temporaneamente un lavoratore, se cambiate nella sostanza la manovra affinché, per esempio, le risorse ricavate siano destinate agli investimenti e alle infrastrutture, specialmente nel Sud, allora ci possiamo ritrovare, ancorché rimanga

a misure elettoralistiche, perché il vostro obiettivo sono esclusivamente le elezioni europee. Questo non è un Governo del cambiamento, è un Governo di natura elettoralistica che pensa di avere - voi stessi pensate - un tempo così breve

che la manovra è troppo debole per dare una spinta all'economia; aggiungo: troppo debole per dare una spinta all'economia che si è già arrestata, che è già in recessione a fronte del probabile arresto dell'economia europea e mondiale.

al Governo? Il Governo ci sta a sentire? Recepisce? Se sì, mi fa piacere, dato che ho una particolare simpatia per il sottosegretario Bitonci, perché è stato anche sindaco. Sono rivolti ai colleghi, di maggioranza o di opposizione? Ai giornali? Per andare sui giornali bisogna sparare delle cavolate enormi!

mi lascia massima libertà di espressione di idee su qualsiasi argomento; non ricevo ordini sul telefonino; sono vicino a Silvio Berlusconi, che in queste ore sta aspettando una sentenza che doveva arrivare da anni. FI-BP)*. Il decreto fiscale è l'aperitivo della legge di bilancio e nella legge di bilancio o nel decreto fiscale, a mio avviso, va fatto un accenno al debito pubblico, che è il problema dei problemi e magari pensare che il condono - chiamiamolo come vogliamo, fatto o non fatto, un'intenzione che pare ritirata - non poteva servire a intaccare il debito pubblico assieme ad altre misure, di cui parleremo in occasione della legge di bilancio. In materia fiscale, come già detto da qualche collega e come abbiamo detto in Commissione finanze, mi pare che non abbiamo fatto semplificazione: abbiamo continuato ad aggiungere norme, che sono arrivate fino all'ultimo momento. C'è un po' di tutto, ma è tranquillamente come tutti i decreti-legge della storia e di tutti i Governi. C'è un po' di tutto dentro; non c'è ordine; non c'è un'idea di un testo unico fiscale o di un riordino che veramente semplifichi la vita ai cittadini. Il condono, a mio avviso, è trattato in modo ipocrita, tant'è che non si usa neanche la parola «condono», Gruppo FI-BP)*. Probabilmente è una questione di ragion di Stato all'interno della maggioranza e le poche cose che erano vero condono sono state rimosse *in extremis*. Il 17 luglio, intervenendo in quest'Aula, avevo detto che, secondo me, per il condono si può abbandonare l'ipocrisia e togliersi ogni remora morale se è finalizzato agli investimenti. corrisponde al detto «Pochi, maledetti e subito» e finanzia la spesa corrente, in realtà intacca il tesoretto che c'è, perché il condono fa parte del monte dei depositi sotto forme diverse, degli italiani, che viene spostato per finanziare la spesa corrente, perché il bilancio dello Stato ha delle spese correnti correnti tutte legittime, ma alcune politicamente giuste e condivisibili e altre meno, come il famoso reddito di cittadinanza. aspettative di gettito, a mio avviso, sono sopravvalutate. Non ci saranno, ma lo Stato, a differenza di un'impresa privata o di un ente pubblico locale, può dire tranquillamente che aspettava un incasso di milioni o miliardi e poi, se questo non c'è, tutto va nel debito pubblico e torniamo donde eravamo partiti. Ma si parla di lotta all'evasione, che va fatta attraverso il condono: in questo modo emerge il reddito non dichiarato e le irregolarità formali, e queste ci stanno.

Noi di Forza Italia obbediamo a un altro principio: gli italiani sono tutti brava gente; tutto è permesso, tranne ciò che è vietato e non il contrario; se c'è qualcosa che non va, ci sono gli organi preposti a controllare e se potessero farlo, lasciando perdere le irregolarità formali, le piccole questioni o i piccoli evasori, forse neanche avremmo bisogno di pensare al condono. Tutto è soggetto a controllo, tutto è ANAC e

spero che il Garante della *privacy* faccia desistere quelli che sono fissati su quest'argomento. Ne ha parlato il collega Damiani la settimana scorsa, al *question time*, e il ministro Tria ha detto che si inventa la fattura elettronica, che sarà applicata, perché le ditte hanno difficoltà a gestire le fatture. Ma dove vive? Le ditte di fatture ne fanno di giorno e di notte, finché vogliono, a miliardi; basta avere la materia per fare una fattura, ossia la vendita di un prodotto o di un servizio. Si fanno tranquillamente. Sono fisicamente contrario alla fattura elettronica - e lo stesso discorso vale per le BCC - perché, a forza di deroghe ed esclusioni, ha creato un altro caos.

Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, il decreto-legge fiscale, dopo varie vicissitudini, approda oggi all'esame dell'Assemblea. Permettetemi di fare chiarezza e di enunciare i punti di forza di questo provvedimento, che contiene importanti elementi, volti a ripristinare un rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato. Contrariamente a quanto espresso in maniera impropria e strumentale dall'opposizione, al fine di screditare l'intero provvedimento, in esso è esclusa ogni finalità condonistica. Il decreto-legge è stato pensato allo scopo di venire concretamente incontro alle esigenze dei cittadini, oggi sempre più in difficoltà, e rappresenta il primo passo verso una riscossione finalmente amica dei contribuenti. È opportuno instaurare una pace fiscale tra l'amministrazione e i cittadini, in modo da rimuovere lo squilibrio economico delle obbligazioni assunte e favorire l'estinzione del debito mediante un saldo e uno stralcio dell'importo dovuto, in tutte quelle situazioni eccezionali e involontarie di dimostrata difficoltà economica. A tale proposito, risulta importante sottolineare che l'articolo 4 sancisce, al comma 1, che sono automaticamente annullati i debiti d'importo residuo fino a 1.000 euro. Tale importo sarà calcolato alla data di entrata in vigore del decreto-legge e risulterà comprensivo di capitale, interessi per ritardate iscrizioni a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Stiamo parlando perlopiù di lavoratori autonomi, piccole imprese e singoli cittadini, non di grandi evasori, come falsamente decantato dall'opposizione. Inoltre, si deve evidenziare che l'intera prima parte del provvedimento è improntata alla pacificazione fiscale. Nello specifico, l'articolo 1 introduce la possibilità di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione, pagando l'imposta contestata, con lo sconto di sanzioni e interessi. Pertanto, con tale decreto si ricostruisce un rapporto tra fisco e contribuente, che, contrariamente al passato, sarà basato sulla reciproca fiducia, comprimendo i tempi di definizione dei verbali conseguenti a un'attività istruttoria esterna, non ancora confluita in un atto impositivo. Al tempo stesso, questo atto provvede ad una semplificazione della gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria. Il concetto di reciproca fiducia è centrale anche nell'articolo 2, il quale introduce la possibilità di definire in via agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli accertamenti con adesione dell'Agenzia delle entrate, in modo da consentire ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali pendenti, ma non ancora definite, versando esclusivamente le sole imposte, senza applicazione delle relative sanzioni e degli interessi. Con l'articolo 3, invece, il debitore potrà beneficiare dell'abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e dell'interesse di mora, come nelle due precedenti rottamazioni, spalmandole in un arco temporale più ampio e con interessi ridotti al 2 per cento. Si crea quindi una nuova idea di fisco, non più oppressore, ma un fisco e uno Stato che si trovano finalmente dalla parte dei cittadini. Emerge, nella conversione del decreto-legge, come prorompente elemento di novità l'articolo 6, che consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, avvisi di accertamento, provvedimenti di erogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione. Le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado, e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Concludo, signor Presidente, ricordando ai colleghi che gli anni di perdurante crisi economica hanno colpito a migliaia gli artigiani, i piccoli imprenditori e i giovani professionisti. Parliamo di cittadini che hanno lottato contro tutto e tutti e che, pur di andare avanti, pagare i propri dipendenti e fare impresa, talvolta hanno contratto debiti nei confronti del fisco. La classe politica si trova nella difficile posizione di dare risposta a queste persone, che ci hanno mostrato le loro difficoltà, le loro paure e l'esigenza di non essere abbandonati dallo Stato. Ci hanno chiesto aiuto e non possiamo voltare lo sguardo da un'altra parte. fiscale è un provvedimento che permette di ridare dignità a queste persone, che permette loro di ripartire e di guardare con speranza al futuro; esso permette di dare sollievo a migliaia di famiglie che hanno lottato contro la crisi e che non si sono arrese. È ora di ripartire tutti insieme. Il presupposto per dare la possibilità a questi cittadini di ricominciare è un fisco amico, un fisco che possa stare dalla loro parte, un fisco che non sia né tiranno, né oppressore, ma che abbia a cuore, accanto alla riscossione dei tributi, anche la possibilità di creare ricchezza e consumi e quindi di contribuire al benessere e alla crescita del Paese.

Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, il decreto-legge che stiamo discutendo contiene importanti misure di carattere fiscale, che vanno nella direzione di andare incontro a quegli imprenditori gravati della crisi economica e in difficoltà nel rispettare i pagamenti delle cartelle esattoriali. Nelle discussioni in Commissione ho verificato come, da parte di alcuni colleghi, ci sia una visione dei contribuenti quali soggetti da perseguire con norme sempre più severe, poiché il contribuente cercherà sempre e sempre più di evadere e frodare il fisco. Io sono convinto che la maggior parte dei contribuenti italiani avrebbe un atteggiamento diverso nei confronti di un fisco più corretto e onesto, insomma un fisco vicino e comprensivo delle difficoltà che si possono manifestare nella vita contributiva di ciascuno di noi. Negli ultimi anni si è andati sempre più appesantendo e complicando il complesso delle norme tributarie, ottenendo pessimi risultati, che ci parlano in maniera inequivocabile di bilanci chiusi civilmente in perdita a causa della crisi economica, con i contribuenti che si ritrovano poi, per effetto di varie riprese e norme di indeducibilità dei costi, con un risultato fiscale positivo, trovandosi però nelle condizioni di non riuscire a pagare le tasse; e tutto questo non per loro volontà, ma per esigenza. Non parliamo poi di quei soggetti che hanno lavorato e prodotto reddito, ma che si ritrovano tra i clienti lo Stato o altri enti pubblici che non corrispondono loro il dovuto nei termini concordati. Questa situazione, dunque, e questo tipo di rapporto vanno cambiati; questa è la direzione che noi vogliamo portare avanti. La rigidità di bilancio a cui questa Europa vuole inchiodare l'Italia ci impedisce di andare immediatamente incontro alle istanze dei cittadini italiani, che, premiando le due forze al Governo, hanno manifestato sensibilmente e chiaramente una volontà di cambiamento che si riflette anche sotto questo aspetto. nostro esame insiste verso questa direzione. Il decreto-legge affronta anche la riforma delle banche popolari, perpetrata dai precedenti Governi, necessaria per accogliere l'istanza di soci delle popolari che si sono visti imporre una riforma senza che fosse loro permesso di poter esercitare il diritto di recesso. Il provvedimento che intendiamo approvare affronta anche la riforma delle casse rurali.

e di cui beneficerà anche il nostro sistema sanitario. Un minor numero di patologie legate al consumo di sigarette significa difatti meno malati a carico del servizio sanitario. al nostro esame, poi, abbiamo voluto introdurre una tassa dell'1,5 per cento nei confronti delle rimesse all'estero fatte dall'Italia verso Paesi extraeuropei, perché ci sembra giusto che chi invia all'estero somme guadagnate in Italia possa contribuire in minima parte alla contribuzione e alla tassazione del Paese che lo ha aiutato a creare questo flusso di risorse. Questo decreto-legge non affronta, però, solo aspetti fiscali, apparentemente freddi e lontani dai cittadini. Fornisce risposte chiare ad esigenze del territorio e della famiglia. Bene quindi il *bonus* bebè a favore di chi ha o adotta un figlio, provvedimento da noi voluto per fornire una misura di contrasto al decremento demografico in atto in Italia, dando quindi un segnale oggettivo. Altro passo importante è l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo in grado di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre dell'anno scorso. Questo fondo, che ha una dotazione iniziale di 476 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, è un indirizzo chiaro nei confronti delle comunità colpite. Quindi, dopo il cosiddetto decreto Genova, ecco un altro esempio di immediata attenzione che questo Governo ha verso le terre colpite da eventi atmosferici catastrofici, tanto imprevedibili quanto insopportabili, e verso quei cittadini che tutto hanno perso. Noi non ci dimenticheremo di loro. Questo decreto ne è la riprova e la conferma.

e assente durante la discussione generale su un decreto-legge che coinvolgerà pesantemente il destino dei nostri concittadini. Detto questo, voglio rimarcare, come hanno fatto anche i colleghi del Gruppo che mi hanno

ed è un settore portante dell'economia nazionale. I prodotti agricoli nazionali di eccellenza sono quelli che nel mondo portano avanti il marchio del *made in Italy*, sono quelli che nel mondo fanno conoscere la nostra specialità

minori rispetto agli ultimi sette anni e soprattutto mi riferisco a quel metodo di redistribuzione di tali risorse che ci saranno nei Paesi membri, che penalizzeranno ancora di più il nostro Paese.

Fratelli d'Italia ha presentato una serie di emendamenti nel merito, per cercare proprio di andare incontro alle esigenze degli agricoltori. Abbiamo presentato degli emendamenti per avere un credito di imposta in agricoltura per le aziende che investono in nuova tecnologia, per un minore consumo del suolo, per un minore inquinamento e per un minore consumo dell'acqua. Abbiamo presentato emendamenti per l'agevolazione delle imposte municipali alle imprese agricole,

Non per ultimo, abbiamo presentato un emendamento che riguarda la sospensione delle multe per le quote latte per l'anno 2014-2015.

nel Consiglio regionale della Lombardia a maggioranza e con un solo voto contrario, in cui il Consiglio regionale chiedeva al Governo di sospendere queste multe, che sono già state all'ente di riscossione e che quindi mettono a rischio la sopravvivenza di tante aziende. Se ne chiede la sospensione semplicemente perché c'è il ragionevole dubbio che queste multe siano calcolate su parametri sbagliati. Infatti, in base anche all'anagrafe nazionale bovina 2014-2015 non c'erano infatti animali da latte sufficienti per produrre quella quantità di latte e quindi

cosa direte alle vostre aziende che producono latte e che rischiano di chiudere, in Lombardia, dove si produce circa il 50 per cento del latte nazionale? Cosa direte ai vostri consiglieri regionali, che hanno chiesto questa sospensione, che oggi qui, invece, respingete? Ebbene, in tutto questo vediamo un Governo del cambiamento che in realtà non ha cambiato nessun metodo, ma ha cambiato soltanto le persone che sono sulle poltrone per decidere. *(Applausi

il decreto-legge sulla pace fiscale, che non è un condono fiscale, contiene numerosi punti che cercano di riconciliare i cittadini contribuenti con un fisco rapace e vessatorio, che ha accumulato un magazzino fiscale di oltre 800 miliardi di euro di crediti fiscali affidati all'Agenzia delle entrate, la cui azione di recupero, sulla quale molti soggetti lucrano, è pari a meno di 50 miliardi di euro. Rispetto al testo originario, lungamente discusso in Commissione finanze e tesoro, sono state apportate numerose modifiche anche per il lavoro dell'opposizione, che dopo l'iniziale ostruzionismo ha scelto una posizione più costruttiva: penso alla riduzione delle sanzioni per coloro che firmano assegni in bianco, ovvero che non contengono nome e cognome del beneficiario e la cosiddetta clausola di non trasferibilità, che aveva suscitato numerose proteste degli incolpevoli cittadini. cittadini. Si cambia anche quella multa minima per gli assegni sotto i 30.000 euro, pari al 10 per cento del valore dell'importo, oltre a sanzioni minori per i piccoli assegni che, al di là dell'importo, andavano da 3.000 a 50.000 euro. Viene cancellato il condono fiscale. viene cancellato! Esso prevedeva che, attraverso la dichiarazione integrativa speciale, si potesse sanare una cifra fino a 100.000 euro. Al suo posto arriva la sanatoria sugli errori formali, commessi fino al 24 ottobre 2018. Poi ci sono altre misure: per esempio, quella per i terremotati: la dotazione fino a 524,6 milioni di

Vi sono altri provvedimenti, per esempio, la deroga alle procedure per la consulenza di investimento del testo unico bancario per l'acquisto di azioni di banche banche di credito cooperativo e banche etiche fino a un massimo di mille euro, che salgono a 2.500 nel caso esista una quota minima per diventare socio superiore a mille euro.

sono poi altri provvedimenti ed uno che sta particolarmente a cuore riguarda l'emendamento che proroga di un anno la trasformazione delle banche popolari dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha rimesso alla Corte di giustizia europea il provvedimento nefasto del Governo precedente:

che prevede una soglia di attivi di otto miliardi oltre la quale una banca popolare deve trasformarsi in SpA. L'ordinanza fa riferimento anche alla circolare della Banca d'Italia che ha disciplinato la materia e, in particolare, al controverso aspetto della limitazione del rimborso del diritto di recesso, che, in base al documento di regolazione, può essere anche azzerato con un rinvio *sine die* del diritto. E guardate che quelle motivazioni del Consiglio di Stato sono una pietra miliare anche di queste autorità vigilanti che stanno sempre dalla parte dei vigilati, e sono possedute dalle banche socie, perché la circolare della Banca d'Italia prevede la possibilità di concedere o negare il rimborso per il diritto di recesso. Infine, signor Presidente, colleghi, mi avvio alla conclusione annunciando che abbiamo sottoscritto l'ordine del giorno del senatore De Bertoldi sulle banche di credito cooperativo, che impegna il Governo a salvaguardare il valore di banche che operano sul territorio, non in base agli algoritmi di Francoforte della Banca centrale europea. di ribadire che provvedimenti, che vorrei definire semplicemente sciagurati, volevano gettarci nelle fauci del *far west* del mercato del *far west* del mercato e della globalizzazione, secondo quella ideologia del neoliberismo dittatoriale, il sacro *Moloch* delle globalizzazioni. La globalizzazione della povertà,

e sulla vita reale di uomini e donne, che ha devastato princìpi e valori costituzionali che noi siamo impegnati a tutelare. Questo non è un condono fiscale: lo ripeto per l'ultima volta!

UV))*. Signor Presidente, l'obiettivo di questo provvedimento era quello di costruire un rapporto più equilibrato tra cittadini e fisco e di favorire un maggior gettito fiscale. Per come giunge in quest'Aula, temo che tante delle misure contenute in questo documento risultino poco efficaci. Ci si è limitati a interventi circoscritti, in alcuni casi di dettaglio, che non si possono configurare come una nuova stagione nel rapporto tra fisco e cittadini. In questo decreto-legge ci sono, tuttavia, diverse misure che riguardano il Sud Tirolo e il Trentino. Vi è lo stanziamento di oltre 500 milioni di euro per i danni del maltempo delle scorse settimane. Le nostre due Province sono state duramente colpite. L'aver stanziato risorse già con questo provvedimento è sicuramente un fatto positivo: lo è per le imprese, le attività commerciali, le famiglie e tutti coloro che, anche nella nostra Regione, stanno vivendo giornate complicate. Vi è la norma che riguarda il credito cooperativo nella Provincia autonoma di Bolzano, e ringrazio al riguardo *in primis* il presidente della Commissione finanze Bagnai e tutti i componenti della Commissione, di maggioranza e di minoranza, che hanno voluto ascoltare le nostre idee e che hanno recepito le richieste del nostro territorio, di cui noi ci siamo fatti portavoce. Con l'emendamento approvato in Commissione, le Raiffeisen, il credito cooperativo nella nostra Provincia, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, potranno optare per un sistema di tutela istituzionale sul modello tedesco, ossia un accordo contrattuale per garantire la liquidità e la solvibilità delle banche partecipanti alla gestione delle crisi, attraverso fondi alimentati dalle banche stesse. Il nostro credito cooperativo è un sistema sano; le nostre banche del credito cooperativo sono solvibili, quindi dare loro la possibilità di non sottostare a una SpA, quindi di aprirsi a un'altra filosofia bancaria, penso sia un un atteggiamento giusto dell'attuale maggioranza. È un modello che ha il pregio di garantire l'autonomia delle banche, di costruire un vincolo di responsabilità rispetto alla tenuta del sistema e, soprattutto, di mantenere quel rapporto con il territorio che è il principio fondativo del credito cooperativo, che lo caratterizza e lo distingue da altre forme bancarie. Vi è, infine, la norma sulla clausola di salvaguardia. Ci tengo a evidenziarla per quanto accaduto con il decreto sicurezza, quando in Commissione l'emendamento fu addirittura dichiarato inammissibile. Questa volta le prerogative delle autonomie speciali hanno avuto la tutela che spetta loro; ed è un bene, perché dovrebbe sempre accadere così. Allo stesso modo, più in generale, ci sono misure che consolidano interventi già sviluppati nella precedente legislatura. Penso alla rottamazione delle cartelle e a tutti gli altri interventi volti a costruire un rapporto più equilibrato col fisco. Penso all'intervento a favore delle partite IVA, su cui già nella scorsa legislatura c'era stato un primo significativo intervento, che con questo decreto-legge ne esce irrobustito. È un bene che siano state confermate le misure a favore delle famiglie, in particolare delle giovani coppie con figli. Ad ogni modo, questo provvedimento deve essere valutato nella cornice complessiva della manovra economica. In più occasioni, anche in quest'Aula, il nostro Gruppo ha espresso le sue perplessità. Non ci convince l'idea di un nuovo indebitamento, lo scontro con l'Europa, a non convincerci sono soprattutto le misure che verranno finanziate. Il reddito di cittadinanza è una misura passiva, che non aiuterà le persone a trovare un lavoro. Non sarà sufficiente la riforma dei centri per l'impiego. L'ho già detto in altre occasioni: i centri per l'impiego hanno difficoltà a funzionare persino in altre

Il lavoro lo creano le imprese, non i decreti o i centri per l'impiego. Le risorse pubbliche devono essere investite per creare sviluppo, per diminuire il costo del lavoro, per stimolare l'innovazione, per migliorare la produttività e la competitività delle imprese. Ben allora, le richieste di correttivi che sta chiedendo anche l'Europa. Soprattutto, ben venga l'atteggiamento dialogante che sta emergendo, dopo l'imbarazzante stagione delle offese all'Europa e dell'isolazionismo dell'Italia. Sarebbe una novità positiva se almeno 3 miliardi venissero spostati sul fronte degli investimenti. Sarebbe un atto di responsabilità, perché siamo in un passaggio delicatissimo: Bankitalia ha calcolato che, dall'inizio della legislatura, gli interessi sul nostro debito sono saliti di 1,5 miliardi per quest'anno, di 5 per il 2019, di 9 per il 2020. L'aumento dello *spread* - come ha ammesso anche il Ministro dell'economia - avrà come conseguenza un aumento del costo dei mutui; inoltre, il *flop* dei BTP italiani, con appena 2 o 3 miliardi prestati dai risparmiatori allo Stato, ci dice tanto sul clima di paura e incertezza che comincia a serpeggiare. Anche per questo bisogna scongiurare in ogni modo le sanzioni europee sulla manovra e puntare con decisione sulla crescita e, quindi, sulla fiducia. In conclusione, signor Presidente, per il tessuto produttivo, per i professionisti dei territori che rappresentiamo, nel provvedimento in discussione ci sono misure positive, ma queste sono insufficienti o inefficaci se non si corregge il tiro della manovra. Il mio auspicio è il seguente:

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, purtroppo - come è avvenuto molto spesso fino ad ora il titolo del provvedimento in esame tradisce sostanzialmente il suo contenuto, perché siamo al cospetto di un provvedimento *omnibus,* nel quale manca una visione di riforma reale del fisco, che è la cosa di cui gli italiani hanno realmente bisogno, visto che siamo il Paese in cui i cittadini pagano più tasse per avere uno Stato più nemico. In questo quadro, il minicondono che viene proposto certamente non rappresenta un'occasione per sanare anche in maniera definitiva le discriminazioni fiscali esistenti. La fatturazione elettronica, inoltre, non è certamente uno strumento per combattere l'evasione, ma rappresenta l'ultima disgrazia per tantissimi piccoli artigiani e piccoli imprenditori che già hanno enormi difficoltà a portare avanti la propria attività e che avrebbero bisogno di strumenti che facilitino la loro professione. Nonostante queste considerazioni,

emendamenti che non propongono la possibilità di nuove tasse, ma che al tempo stesso aiutano i Comuni a far quadrare

servizi e risposte per i cittadini, Fratelli d'Italia ritiene giusto sostenere. Per questo motivo noi auspichiamo che il contributo che viene dal nostro Gruppo possa rappresentare quella manina buona che dà agli italiani un'occasione di sollievo rispetto alle misure assolutamente insufficienti del decreto-legge Signor Presidente, per quanto riguarda la posizione generale che il Partito Democratico assume verso il in esame, penso che la relazione di minoranza del senatore d'Alfonso sia stata esauriente, articolata, incisiva e motivata punto per punto, per il lavoro che è stato fatto in Commissione. Il Partito

In particolare, mi vorrei soffermare sul tema dell'edilizia convenzionata e agevolata. La proposta di modifica approvata dalla maggioranza in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi costruiti in edilizia convenzionata e agevolata affronta il problema, ma solo limitatamente. La disciplina dell'edilizia convenzionata ha subìto nel corso del tempo una continua evoluzione attraverso numerosi interventi legislativi. Tuttavia, credo che si imponga oggi una modifica organica e omogenea della normativa di riferimento, considerando che l'attuale situazione dei piani di zona realizzati in regime di edilizia agevolata necessita di interventi normativi urgenti per risolvere alcune criticità del sistema, a tutela di tutti i soggetti interessati. Coerentemente a questa impostazione, abbiamo presentato un emendamento che intende ribadire la funzione economico-sociale che ha ispirato il legislatore nei tempi passati nella materia dell'edilizia convenzionata e agevolata. L'emendamento in questione marca in maniera determinante l'intero impianto normativo, assicurando il bene primario «casa» a categorie di soggetti ritenuti svantaggiati in quanto privi della potenzialità economica per entrare nel libero mercato immobiliare. La suddetta proposta ha il fine di razionalizzare in modo uniforme e trasparente i procedimenti di trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà e di rimuovere i vincoli relativi alla commerciabilità e ai prezzi di alienazione e locazione. Viene favorito altresì il completamento dei piani di zona, prevedendo la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Infine, viene introdotta una disciplina volta a risolvere in via definitiva le questioni insorte tra venditori e acquirenti degli alloggi per la violazione delle convenzioni relativamente alle norme in tema di prezzo massimo di cessione, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme di legge. In particolare, l'emendamento da noi proposto prevede la possibilità per i titolari del diritto di superficie di richiederne la trasformazione in diritto di proprietà, obbligando i Comuni a individuare le aree non soggette a trasformazione e a rispondere alle richieste dei cittadini entro un termine certo, oltre il quale scatta il silenzio-assenso. Viene stabilito un procedimento per la determinazione del valore venale delle aree, caratterizzato da certezza e oggettività, in quanto riferito ai rilevamenti dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Un ulteriore aspetto affrontato dalla nostra proposta riguarda la parità di trattamento giuridico tra i titolari di convenzioni, aventi a oggetto il diritto di proprietà piena, e coloro che hanno ottenuto la stessa piena proprietà a seguito della trasformazione del diritto di superficie, attraverso la decadenza di tutti i vincoli alterni dei vent'anni a partire dalla data di stipula della convenzione originaria. Dunque, i vincoli eliminati non sono solo quelli relativi al prezzo massimo di cessione, come invece avviene con l'emendamento approvato dalla Commissione e proposto dalla maggioranza. Infine, tutti i corrispettivi acquisiti dai Comuni in seguito alla cessione delle aree conseguenti alla trasformazione saranno destinati al completamento di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona, anche nell'ottica di ristabilire i principi di legalità e sicurezza per i cittadini. Invito i colleghi della maggioranza a tenere in considerazione l'approvazione di quella proposta emendativa, che è organica, attraverso la quale sarà possibile tracciare una linea di discontinuità con l'esperienza passata che permetta di risolvere molte delle problematiche attualmente esistenti e rilanciare il comparto dell'edilizia residenziale pubblica, come risposta

- intervengono su alcune emergenze. Quindi, ben venga che ci sia un fondo di 500 milioni di euro per il solo anno 2019 e altri 50 milioni di euro per l'anno successivo, finalizzati in particolare al settore di spesa dell'edilizia pubblica, ivi comprese la manutenzione e la sicurezza, nonché la manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico

si è riproposto un provvedimento che viene dal passato e che il Governo ha deciso di rifinanziare. Sto parlando del *bonus* bebè,

alla natalità. In un Paese - è risaputo - vecchio come l'Italia, bisogna mettere in campo

garantire loro un futuro. Do solo qualche dato, perché la forza dei numeri è sempre potente. La popolazione anziana, sopra i sessantacinque anni, al 1° gennaio 2018, conta 13.644.363 persone e rappresenta il 22,55 per cento della popolazione totale italiana.

implica tante altre cose: quante pensioni dovranno essere pagate, quali sono le fasce che invece dovranno lavorare per pagare le pensioni. È un dato davvero importante, per cui occorre che vengano messe in atto tutte quelle proposte per far sì che il tasso di natalità aumenti

che ha destato grandissima preoccupazione in tutta la zona al confine con la Svizzera: il Governo ha optato per la nomina di un commissario straordinario, incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco, che si dovrà raccordare con gli enti locali, territoriali e non, della Lombardia.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, cittadini che ci seguite attraverso la televisione e i canali *social,* al nostro esame interveniamo per cominciare a risolvere alcune criticità del nostro sistema tributario. Veniamo incontro alle persone e ai cittadini che si sono trovati in difficoltà con il fisco a causa della crisi devastante che ormai da più di un decennio prosciuga le risorse più importanti del nostro Paese. Interveniamo sulle criticità di un sistema tributario che ha una pressione sui cittadini ormai insostenibile a causa degli spaventosi livelli dell'evasione fiscale, che non trova eguali non solo in Europa, ma - credo - in tutti i Paesi dell'Occidente sviluppato. Abbiamo un numero di cittadini che purtroppo continua a sottrarsi al patto sociale che sottintende ed è sottoscritto nella nostra Costituzione.

stremati anche per i vincoli che ci derivano dagli obblighi di servire un debito pubblico che costa ogni anno ai cittadini la bellezza di circa 65 miliardi. Pensate: 65 miliardi di euro l'anno di interessi causati da decine di anni di politiche economiche che sono servite, il più delle volte, alle nostre classi dirigenti per sperperare risorse preziose nel nome di politiche che tendevano a gestioni clientelari, elettorali e fondate sugli sprechi. È la politica economica che ha unito Governi di centrodestra e di centrosinistra e ha fatto schizzare il nostro debito pubblico oltre i 2.000 miliardi, cifre che ben conoscete e che sono note al Paese, che rappresentano oltre il 130 lordo. Al Paese, stremato e preoccupato, noi veniamo incontro con le misure che vi sono state elencate questa mattina e che vanno dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione fatti ai contribuenti, alla definizione agevolata degli atti di accertamento, alle cancellazioni delle cartelle esattoriali

quella massa immensa di ruoli, pari a 850 miliardi di tasse non riscosse che, a causa degli scandali degli enti di riscossione, privati cittadini, spesso mafiosi, banche che hanno truffato, hanno reso impossibile, alla fine di un faraginoso e difficoltoso processo di accertamento e contestazione delle delle cartelle agli evasori, persino mettere le mani alle risorse certe che un sistema fiscale ingiusto e inefficiente, pur tuttavia in capo anche a decine di anni di lavoro, era riuscito a definire rispetto agli evasori fiscali. Ci sono altri temi importanti sui quali interveniamo che si accostano alla tematica fiscale, ma che riguardano altre priorità del nostro Paese; misure apparentemente di poco rilievo - se volete - rispetto alla massa dei nostri problemi, come aver previsto l'incompatibilità tra il ruolo di Presidente di Regione e quello di Commissario straordinario ai piani di rientro, che spesso ha significato una gestione più attenta agli interessi elettorali

in radice un conflitto di interessi che - voglio ricordarlo per i Presidenti di Regione in Aula - negli ultimi dieci anni ha significato spesso avere senatori incompatibili. È, infatti, ancora possibile eleggere senatori consiglieri regionali e Presidenti per i quali la nostra Costituzione prevede l'incompatibilità. Preannuncio che interverremo interverremo sull'articolo della Costituzione che tratta il tema per rendere questa incompatibilità una stringente e chiara causa di ineleggibilità.

primaria della rete di telecomunicazioni, che tanti soldi era costata ai cittadini, a un prezzo vile a privati che poi l'hanno saccheggiata.

rispetto alla tutela delle infrastrutture pubbliche e strategiche per il Paese, offriamo la possibilità di sanare uno scandalo e una gestione folle, riportando in capo alla proprietà pubblica la rete delle telecomunicazioni, che sarà cruciale per garantire a tutti i cittadini nei prossimi anni quell'accesso adeguato e veloce a Internet che la modernità richiede. Questi sono

idrogeologica. E il decreto trova risorse per dare ai cittadini ciò che ci stanno chiedendo pagando fino in fondo ogni anno le loro tasse. Per questo lasciatemelo dire - risultano incomprensibili le critiche delle opposizioni al provvedimento, a cominciare da quelle del Partito Democratico. Sono misure che i cittadini ci chiedono e che avrebbero meritato, dal mio punto di vista, un'attenzione maggiore

il futuro del nostro Paese e delle giovani generazioni. È il nodo scorsoio del debito pubblico. I cittadini italiani, a partire dal 1980, hanno pagato circa il doppio del debito pubblico. Dobbiamo intervenire per trovare risorse, per sanare e togliere dall'Italia questo peso immenso che - il futuro delle nuove generazioni. E lo possiamo fare espandendo l'economia: ci proviamo e ci abbiamo già provato, trovando le risorse per fare gli investimenti necessari, ma lo dobbiamo fare andando a pescare

ma soprattutto trovare le risorse per finanziare la speranza e lo sviluppo del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo

torturare i contribuenti emersi, che, pur potendo sbagliare, dichiarano e sono tracciabili e rintracciabili dal fisco. Non è questo il rapporto che vogliamo per creare entrate. Vogliamo che l'obiettivo sia ricreare un virtuoso rapporto tra fisco e contribuente, che semplifichi quindi la vita alla spina dorsale del Paese, cioè agli imprenditori e ai professionisti, e che lasci loro fare ciò a cui sono preposti, ossia creare beni, servizi e posti di lavoro. Non serve a niente il reddito di cittadinanza, se si impedisce alle imprese di creare posti di lavoro. Lo Stato, quando introduce obblighi a carico dei contribuenti, deve porsi prima il problema di essere esso stesso *compliant*.

a chiedere a carico dei contribuenti obblighi che dovrebbero gravare a carico dello Stato? Non è questo il diritto, ma è uno Stato civile quello che vogliamo. Se si introduce la fatturazione elettronica, non si può nemmeno pretendere che l'onere di archiviare tutta la documentazione sia a carico e a costo dei contribuenti, che devono acquistarsi i *software*

hanno le loro difficoltà a tenere l'Italia a galla in un mercato globale e complicato. Stiamo affossando il Paese, non gli stiamo dando la spinta per crescere.

L'obiettivo del decreto fiscale - sembrerà banale dirlo - è occuparsi della materia fiscale. Sotto questo profilo, non abbiamo assolutamente capito perché sia diventato un *pot pourri*, un *omnibus* di materie assolutamente importanti. Si è rischiato di destabilizzare settori fondanti del nostro Abbiamo evitato il peggio e abbiamo vigilato, affinché settori strategici, come quello che rappresenta l'11 per cento del credito, quale il credito cooperativo, non venissero smontati per decreto a pochissimi giorni dall'entrata in vigore della riforma. Abbiamo spinto per trovare una soluzione al contenzioso sul prezzo massimo di cessione innescato dalla sentenza n. 18135 della Cassazione a sezioni unite. Abbiamo lottato come sempre per i balneari, per lo sport per quello dilettantistico. Abbiamo evitato che le autostrade diventassero ostaggio del nuovo nazionalismo del Governo. Abbiamo vigilato e vigileremo affinché l'idea di rete unica, che pure ha in sé dei tratti di positività, non diventi terreno di monopolio delle informazioni, rischiosissimo in uno Stato democratico Continueremo a vigilare, perché noi vogliamo portare l'Italia di nuovo in Europa; vogliamo portare l'Italia di nuovo ai vertici della produttività, del bel pensiero, del bel futuro.

io mi pongo anche una domanda sul valore e sul significato della replica, quando la replica spetti al relatore di maggioranza, quando la replica spetti al relatore di minoranza. E sono convinto che la replica non sia una coda, indebolita tematicamente, della parte inizialmente espressa. La replica si nutre dei punti di vista ascoltati ed è l'ultimo, estremo tentativo di chiamare a ragionevolezza e a riflessione Io con questo spirito contribuisco alla ragionevolezza di quest'Aula, tenendo da conto tutti gli interventi che ci sono stati. stati. L'ordinamento tributario è messo al riparo da uno dei principali istituti di democrazia che la nostra Carta prevede, la sottoposizione al *referendum*, perché la materia tributaria - direbbe Norberto Bobbio - è materia sacrale; grazie a questa materia si edifica il costituito della nostra collettività.

produce e mette in campo un costo culturale e morale di diseducazione di cui noi ci dobbiamo fare carico. Io non prevedo una democrazia angelica e senza errori; la democrazia dentro di sé può dare luogo a errori. Il punto è che il confronto dialogico, il contraddittorio, l'ascoltarsi, il dire e l'ascoltarsi poi devono dare luogo alle correzioni. Qual è il problema - per esempio - dello stralcio annullante riguardante le cartelle fino a 1.000 euro di quel decennio? Si può scatenare, in capo al cittadino, la scommessa di attendere un'altra operazione di stralcio. Questo è il punto del quale vi dovete e ci dobbiamo fare carico. Così come sparare operazioni di rottamazione, senza che si sia patrimonializzata dal punto di vista amministrativo la rottamazione precedente, ha con sé un carico infettivo. Noi dobbiamo dare luogo a una condotta fiscale e tributaria che è tipica dello Stato e, non di una liofilizzazione dello Stato o di un ologramma dello Stato. Guardate che tutti gli studiosi e i politici, anche di parti che adesso hanno fatto sentire il proprio il proprio punto di vista, evidenziano che sulla materia tributaria ci vogliono più serietà, meno intermittenza, meno casualità, meno improvvisazione; tant'è tant'è che l'ordinamento normativo prevede, ad un certo punto dell'esercizio legislativo, il decreto-fiscale, per fare in modo che abbia compiutezza e omogeneità di materia, evitando che si trasformi in un'arca sbagliata. corre il rischio di essere un'arca sbagliata. Io mi devo complimentare con pochi, a volte introvabili, ma comunque significativi interlocutori nella Commissione; pochi e a volte introvabili, perché presi da un grande carico di lavoro. Devo riconoscere lo sforzo che ha fatto il sottosegretario al MEF Bitonci, che ha provato più volte a cucire e ricucire un impazzimento di condotta di una coalizione che tirava come l'asino di Buridano, da una parte parte opposta, correndo il rischio di morire di acqua e anche di cibo, perché non c'era, al di là dello scritto, alcun accordo su niente. Detto questo, apprezzo lo sforzo compiuto sull'adempimento collaborativo (un emendamento del PD), che fa in modo di statuire una reciprocità di lealtà collaborativa fiscale: lo Stato e l'imprenditore produttore di ricchezza insieme. Avevamo chiesto un altro emendamento: il cittadino onesto che paga, e paga di più, deve essere rimborsato Non può esserci comprensione per chi non paga, astutamente, e non, invece, disponibilità per chi ha pagato di più. Voglio ringraziare - e concludo quell'attenzione "angelica" che c'è stata sull'emendamento riguardante la defiscalizzazione delle rendite INAIL. È stato compiuto un errore,

fiscale. Abbiamo presentato un emendamento abbiamo e avuto attenzione. Il senatore Bitonci e anche il presidente Bagnai, molte volte soccorso e soccorrente anche con la sua cultura laterale, ci hanno dato attenzione ma, anziché l'emendamento approvato, è venuto in campo un ordine del giorno con la forza della raccomandazione. In Europa, quella che a tratti è odiata, la raccomandazione produce anche norme; mi auguro - e concludo che la curvatura delle intelligenze dia luogo ad un recupero di rettilineo normativo.

Sospendo pertanto la seduta

vorrei stigmatizzare la modalità con la quale stanno procedendo nei nostri lavori. Apprezzo che la Presidenza abbia celermente preso atto del fatto che non siamo ancora nelle condizioni di procedere poiché la Commissione bilancio non ha ultimato i propri lavori. Sicuramente non li ha ultimati in modo ordinato e, quindi, deve mettere in ordine i fascicoli, cosa che ci sta portando ad arrivare in Aula con tre testi in parallelo e ciò renderebbe molto difficile orientarci sia nella valutazione che nell'indicazione di voto

impossibilità di iniziare a votare alle 15,30, fa sì che il Gruppo del Partito Democratico si ritenga libero da qualsiasi accordo preventivo, semplicemente per una questione di rispetto dei lavori e di tutti coloro che siedono in quest'Aula.

Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire.

intanto vorrei ringraziare il presidente Bagnai, tutti i funzionari della 6a Commissione del Senato, ma devo dire soprattutto i commissari, senatori di maggioranza e di opposizione, perché mai come questa volta il testo è stato essenzialmente migliorato - com'è stato ribadito anche prima - grazie a un attento lavoro della Commissione e dei colleghi. Adesso vi farò anche qualche esempio specifico in cui l'attività emendativa ha portato a un miglioramento sostanziale del testo.

è stata espunta anche la dichiarazione integrativa speciale, il testo è diventato una vera e propria pace fiscale. Era infatti nell'intento e nella *ratio* originaria cercare una soluzione in cercare una soluzione in quello che è un rapporto migliorato con il cittadino contribuente. Ed è per quello che dal precontenzioso, passando attraverso le liti pendenti

la *ratio* su cui è stato costruito il provvedimento, che è estremamente ampio rispetto ai precedenti: si va dai primi processi verbali di constatazione, fino ad arrivare all'ultimo grado della Cassazione.

introduce un tema fondamentale, che ritroveremo nel decreto legislativo sulla crisi d'impresa, relativo alla transazione fiscale, cioè alla possibilità di arrivare a una definizione del rapporto tra il cittadino, l'impresa e il contribuente attraverso una verifica dell'effettiva valutazione della situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, uno di quegli adempimenti che già in altri Stati viene utilizzato con grande successo. È per questo che esprimeremo parere favorevole

era un ampliamento totale; noi facciamo un ampliamento parziale, per gradi, sapendo che già nel decreto legislativo sulla crisi d'impresa abbiamo inserito la novità sulla transazione, che ritengo estremamente importante. Un'altra novità importante che ha migliorato il decreto‑legge è stata sicuramente la sanatoria delle irregolarità formali, che ha completamente sostituito la dichiarazione integrativa speciale. Tutti gli errori che vengono fatti nella presentazione della dichiarazione e nella firma

dando un indirizzo preciso su quella che dovrebbe essere l'impostazione del rapporto tra i contribuenti e il fisco e in qualche modo rappresenta una piccola rivoluzione in questi rapporti. L'adempimento collaborativo, infatti, si fonda sul principio dell'affidamento e del reciproco rispetto tra impresa e fisco, con un fisco che vede e controlla dove possono esserci dei problemi, ma anche con un'impresa che vede, suggerisce e chiede al fisco, in maniera preventiva e con tempi certi sugli interpelli, come potersi meglio orientare.

Il contribuente che aderisce all'adempimento collaborativo deve in qualche misura dotarsi di un regime che gli permetta di analizzare, controllare e verificare tutte le proprie scadenze fiscali e può essere esteso a tutti i soggetti che abbiano la capacità di semplificare il rapporto con il fisco nazionale. L'adesione a tale regime fiscale ha l'obiettivo di favorire l'interlocuzione costante e preventiva tra i contribuenti e l'Agenzia delle entrate ed è volta a definire in anticipo, sulla base di elementi di fatto, le obbligazioni tributarie in capo al contribuente. Per tali ragioni crediamo che l'emendamento 01.1 (testo 2) possa dare più sostanza al decreto fiscale che dovrebbe andare a nostro giudizio a modificare in maniera positiva il rapporto tra il contribuente ed il fisco.

ai contribuenti stessi per poter recuperare eventuali somme pagate in eccesso. Il decreto-legge, così come confezionato dal Governo, si caratterizza per essere un provvedimento che favorisce favorisce il recupero dei ritardi, pagando sanzioni limitate e mettendosi un po' al riparo rispetto a sanzioni che sono sicuramente onerose. Ma nel momento in cui lo Stato consente a un contribuente di poter avere dei benefici su ritardati pagamenti o multe e dà la possibilità di recuperare qualcosa sull'evasione sanzionata, crediamo che sia corretto consentire a quei contribuenti che, invece, hanno che, invece, hanno pagato di più e nei tempi dovuti di richiedere l'equo rimborso in un lasso di tempo uguale a quello al quale si consente a chi ha evaso di poter beneficiare di quanto il decreto prevede. Quindi, la richiesta è quella di prorogare a cinque anni, a sessanta mesi le possibilità di recupero di quanto si è pagato di più. Con questi due emendamenti, che di fatto costituiscono due pre-articoli dell'articolato del decreto stesso, vogliamo dare una una caratterizzazione migliore a questo decreto fiscale che va nella direzione di favorire il rapporto tra il contribuente e il fisco, da un lato,

Presidente, noi ci siamo approcciati al decreto-legge fiscale con una visione diversa da quella che poteva sembrare all'inizio, cioè abbiamo cercato, in ogni passaggio, di distinguere coloro che secondo noi non hanno alcun diritto di partecipare a questa sanatoria e a questo condono da coloro che invece, in linea di principio, avrebbero potuto parteciparvi. L'emendamento 1.17 va appunto nella direzione di distinguere l'evasore incallito da tutto il resto del mondo. Chi è l'evasore incallito? È colui che intende partecipare a questa sanatoria pur avendo partecipato in passato ad altri condoni fiscali, ad esempio. È colui che intende partecipare a questa sanatoria non avendo mai presentato dichiarazione redditi in passato. colui che, nel passato oppure adesso, intende sanare la sua posizione dopo aver evaso almeno la metà del proprio capitale sociale o oltre la metà dei redditi che vorrebbe sanare. Questo signore, che in passato ha già partecipato a condoni, questo signore, che ha dimostrato una volontà evasiva pervicace e continuativa, a nostro modo di vedere non dovrebbe avere diritto a partecipare a null'altro, perché partecipa in maniera attiva e cosciente a deprimere le casse e l'erario dello Stato. Questo signore è recidivo. Pertanto, con il nostro emendamento, chiediamo che sia escluso da questa sanatoria, in modo che vi sia un segnale chiaro da parte dello Stato e dell'erario nei suoi confronti.

ma non hanno poi perfezionato la procedura sanando i debiti che avevano chiesto di sanare. Chiediamo cioè di escludere questo tipo di contribuenti per due ragioni fondamentali, non per avversione nei confronti di questi contribuenti.

perché colui che non lo ha fatto adesso ha un'agevolazione maggiore rispetto a coloro che nello stesso periodo avevano chiesto di partecipare, visto che viene offerta loro una possibilità molto più Il secondo principio che vogliamo tutelare è quello di evitare che lo Stato, nella sua amministrazione fiscale, rimetta sempre in discussione le scelte fatte in passato con regole nuove, che peraltro vanno a incidere su situazioni *in itinere* come quelle che ho descritto. Per queste due ragioni chiediamo che alla rottamazione di cui all'articolo 3 non partecipino coloro che in passato, pur avendone fatto richiesta, non hanno sanato i debiti che avevano chiesto di sanare.

la motivazione di questo emendamento risiede nel fatto che le sanzioni amministrative in materia di lavoro sono talmente sproporzionate rispetto agli eventuali illeciti in cui può incorrere il datore di lavoro nella gestione dei rapporti con il personale dipendente che determinano una vera e propria vessazione nei confronti dei legali amministratori delle aziende, ancorché cessate o fallite, che non possono corrispondere quanto dovuto, con evidente danno per l'amministratore che risponde personalmente con il proprio patrimonio. Un esempio eclatante che tutti ricordano è quello accaduto a un panettiere della Provincia di Napoli, che si tolse la vita per aver ricevuto un verbale dell'ispettorato del lavoro al quale non poteva ottemperare per le ragioni che che ho appena spiegato. Chiedo quindi all'Assemblea di approvare questo emendamento, che peraltro non comporta alcun onere, ha il nulla osta della Commissione bilancio e serve ad estendere le previsioni già contenute nel decreto-legge anche ai rapporti di lavoro per aziende fallite, che oggi sono escluse e non hanno nessuna possibilità di risolvere i problemi nati in questo frangente.

a seguito della cancellazione di quanto previsto dal presente articolo e quindi la possibilità di procedere a un riaccertamento puntuale dei residui al 31 dicembre 2018.

di escludere i tributi delle Regioni, delle Province e dei Comuni dalla trattazione. Infatti, come è stato evidenziato anche dall'analisi in Commissione, la possibilità che lo stralcio dei carichi pendenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, fino a 1.000 euro, abbia un peso rilevante nei bilanci dei Comuni. Questa riflessione è stato oggetto

questo organismo ha posto l'attenzione sul tema dei rimborsi riguardanti le spese per le procedure di riscossione che hanno messo in essere i Comuni. Queste spese non trovano alcun tipo di rimborso e sono a carico degli enti.

sotto due profili, che sono stati posti alla nostra attenzione dall'Associazione nazionale dei Comuni, attraverso l'intervento in Commissione del sindaco Nogarin, quindi attraverso un contributo non di parte ma del tutto istituzionale.

perché la legge interviene direttamente sui crediti degli enti locali, senza prevedere una diretta compensazione. Tra l'altro, si tratta di crediti che potrebbero essere ancora presenti nei bilanci dei Comuni perché considerati esigibili. C'è, poi, un aspetto finanziario, perché questo stralcio stima una possibile perdita nei bilanci dei Comuni per cifre che vanno dai 3 ai 5 miliardi di euro. È pur vero, e vado a concludere, che nel 2015 è intervenuto, attraverso il decreto legislativo n. 118, il riaccertamento straordinario dei residui e quindi molti Comuni, quasi tutti, hanno ordinato i propri bilanci e stralciato da essi i crediti definiti inesigibili. Però, all'interno dei Comuni sono rimasti anche crediti datati, cioè ascrivibili al periodo 2000-2010 perché considerati esigibili; tale aspetto potrebbe determinare

di far sì che si potesse ridurre l'impatto sui bilanci, garantire l'autonomia costituzionale degli enti locali nonché l'equità tra i contribuenti. La nostra proposta voleva soprattutto dare a questi elementi un'attenzione centrale.

quelli che non hanno dichiarato, ci sta molto a cuore dire che forse la rottamazione dei ruoli avrebbe dovuto essere estesa ai contribuenti che sono in grave

l'articolo sulla rottamazione non tiene assolutamente in considerazione il combaciare delle situazioni tra la rottamazione uno e la rottamazione *bis*, creando delle differenziazioni e delle disparità tra contribuenti davvero non accettabili in un ordinamento di Stato civile come il nostro. In termini di raccordo, non si capisce neppure come mai siano presi in considerazione soltanto i ruoli iscritti fino al 31 2017 e non fino all'entrata in vigore del decreto-legge. Erano provvedimenti molto attesi dalla totalità dei nostri cittadini che il Governo non ha ascoltato.

Per quanto riguarda il contenzioso tributario di primo grado si dà luogo al superamento della controversia laddove ci sia stata soccombenza con il riconoscimento di una consistenza finanziaria che fa riferimento al dovuto del contenzioso. Allo stesso modo, c'è una valutazione di questo tipo laddove c'è stata soccombenza al secondo grado. Qual è limite di questa norma per cui ne chiediamo la soppressione? Interviene sulla manifestazione del problema e non sulla causa del problema. Noi in Commissione, dove non abbiamo fatto un lavoro - come ho ripetuto anche questa mattina in due circostanze due circostanze - di arredamento o di abbellimento, abbiamo suggerito di lavorare sulle cause che creano un'eccessiva consistenza numerica e finanziaria di contenzioso tributario di primo e secondo grado. Abbiamo ascoltato dalle rappresentanze della magistratura tributaria questioni riferite al numero delle competenze professionali di cui alla magistratura tributaria, all'attrezzatura tecnologica delle commissioni tributarie di primo e secondo grado e poi abbiamo anche misurato la difficoltà della sede, che atecnicamente posso definire di terzo grado, che è la Cassazione. Ma l'anomalia delle anomalie è che noi, nelle schede di bilancio riguardanti il MEF, troviamo un rimpicciolimento di dotazione finanziaria proprio per il funzionamento delle commissioni tributarie. Non si possono togliere le risorse alle commissioni tributarie, rilevare la loro inefficacia e inefficienza e poi introdurre una norma, in occasione del fiscale, che produce scontistica. È un atteggiamento da Gian Burrasca, perché non si lavora in maniera da potenziare la fisiologia, si genera il meccanismo che produce la patologia e poi si rincorre il problema dell'organizzazione con norme straordinarie. Per questa ragione diciamo: scavalchiamo, superiamo, evitiamo l'articolo 6 e lavoriamo per irrobustire la capacità dell'ordinamento tributario italiano, perché non si tratta di cento o di mille cause, ma si superano le centinaia di migliaia di cause, come stanno gli avvocati e i commercialisti presenti che si occupano di questo. che si occupano di questo. C'è inoltre la genuinità del parere che noi abbiamo acquisito da parte delle associazioni sentite. Per queste ragioni mi auguro che l'Assemblea voglia andare oltre la tristezza dell'articolo 6, per lavorare invece su una dotazione normativa che faccia funzionare l'ordinamento

Signor Presidente, io inviterei il Governo, soprattutto la parte verde del Governo, a riflettere su questo emendamento. Esso infatti non è altro che la traduzione di una promessa fatta dal centrodestra in campagna elettorale. Noi avevamo promesso la pace fiscale non per favorire i furbetti del quartiere, ma per garantire un sistema impositivo che

Questo emendamento, che pone fine a un contenzioso di 21 milioni di procedimenti che non porteranno quasi nulla nelle casse dello Stato, un contenzioso che ammonta a 100 miliardi di euro, potrebbe far ricavare alle casse dello Stato qualcosa come 15-20 miliardi di euro. E allora sì che la *flat tax* potrebbe essere attuata! Mi rivolgo agli amici della Lega: avete ingoiato il reddito di cittadinanza, che sono 10 miliardi di spesa improduttiva, soltanto per consentire ai vostri alleati di Governo E allora un po' di resipiscenza, uno scatto di dignità e di orgoglio: votate questo emendamento e rientrate nel seminato del centrodestra, quello che voi avete sostenuto. Queste sono le promesse che voi avete sottoscritto in campagna elettorale e che avete sottoscritto con tutto il centrodestra.

6.14, 6.15, 6.16 e 6.17.

Molto spesso - come in questo caso - emendamenti proposti dal Gruppo Forza Italia e anche da altri Gruppi sono stati presi in considerazione

decreto-legge - che avrebbe dovuto rasserenare il clima tra il contribuente e l'erario. Era stato presentato con la possibilità da parte dei contribuenti che non avevano subito accertamenti di poter regolarizzare la loro posizione con una denunzia integrativa:

di regolarizzare chi effettivamente aveva una situazione fiscale serena non colpita dall'accertamento. È stata una scelta; ne abbiamo preso atto, ma questa scelta ha avuto naturalmente delle ricadute sull'*iter* del provvedimento perché, come per i contribuenti privati e i soggetti giuridici, si è negata questa possibilità anche alle società sportive dilettantistiche. Parliamo di un mondo che nasce sulla base del volontariato. Parliamo di un mondo che ha avuto, sino ad oggi, una logica di norme tributarie del tutto articolate e contraddittorie l'una nei confronti dell'altra. Sui contenziosi, vorrei fare soltanto dei piccoli cenni per dire ai colleghi come la normativa fiscale relativa alle società dilettantistiche sia stata alquanto controversa ed alquanto pasticciata nel tempo. Per esempio, i funzionari dell'Agenzia delle entrate e i militari della Guardia di finanza hanno spesso dato le interpretazioni più disparate alle leggi, che sono state estremamente complesse. Ad esempio, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 9/E del 24 aprile 2013, ha ritenuto opportuno intervenire per mitigare le pesanti prese di posizione dei propri uffici e della stessa Guardia di finanza. Addirittura, resasi conto delle innumerevoli contestazioni sorte a seguito del fatto che venivano battezzati come sponsorizzazioni molti proventi di pubblicità, che godevano, questi ultimi, ai fini della detrazione forfettaria, di quella del 50 per cento contro quella del 10 dei proventi di sponsorizzazione, la stessa Agenzia ha proposto la norma che prevede la detrazione del cento dei proventi. Cosa voglio dire, colleghi? Si tratta di un terreno dove non vi è stata chiarezza del legislatore e non vi è stata chiarezza, anche interpretativa, da parte dell'Agenzia delle entrate e da parte degli accertatori. che, quindi, ha creato momenti di insicurezza a carico degli stessi dirigenti delle società dilettantistiche. Si dirà, da parte di alcuni, il condono) è diseducativo perché, sostanzialmente, aiuta ad evadere: nel momento in cui c'è il condono, si sana in maniera forfettaria il pregresso e, quindi, si può sperare in un futuro condono e si continua ad evadere. Ma vogliamo applicare questo principio ai dirigenti delle società dilettantistiche, che operano soltanto grazie alla loro buona volontà, per un interesse principale, che è quello di educare i nostri giovani, non soltanto allo sport, ma anche all'educazione civica, al rispetto delle istituzioni e alla sanità del competere? Vogliamo interrogarci? Io voglio dire ai colleghi, e lo voglio dire anche al Governo e alla maggioranza, che qui non si tratta di un'eccezione, ma si tratta di dare un segnale

che non hanno subito accertamenti, che non hanno verifiche, che sono in regola, di poter sanare in maniera definitiva le loro posizioni con un versamento integrativo del 20 per cento dell'Ires e dell'IRAP? Vogliamo dare questo segnale? Io non credo che commetteremo un gesto sbagliato, signor Presidente e colleghi,

tanti giovani, uomini e donne, che hanno portato alto il vessillo della nostra Patria, vincendo medaglie d'oro alle Olimpiadi e ai campionati del mondo, onorando il nostro Paese. Infatti, è dal mondo dilettantistico che è venuto il meglio del nostro Paese, non da quello professionale.

Ogni azienda, fuori da questo Palazzo, si aspettava una risposta da questo Governo, che nasce da due forze politiche e che ha promesso sin da subito di dare risposte al Paese, motivo per il quale due forze diverse, con due programmi completamente differenti, si sono messe insieme. ci aspettavamo, da cittadini prima e da politici poi, una risposta verso le nostre imprese, che stanno soffrendo la crisi ormai da diversi anni. Certo, non ci aspettavamo una vera e propria riforma fiscale, una *flat tax* vera e propria, così come concepita dal programma del centrodestra, ma quantomeno una riduzione delle tasse. Questo non è accaduto,

Signor Presidente, questo emendamento tiene conto della difficoltà che le bande stanno affrontando a seguito della riforma del terzo settore. Abbiamo parlato prima di quanto sia importante investire sui nostri giovani per le attività sportive. Ebbene, credo che le attività culturali, quelle che danno la possibilità ai nostri giovani di esprimersi liberamente e di fare vita sociale,

a una delle ingiustizie più eclatanti che sono contenute nel decreto-legge in esame. I produttori delle cosiddette sigarette elettroniche devono allo Stato 177 milioni di euro di imposte e il fatto che li debbano è stato confermato da una sentenza del TAR e da un successivo intervento della Corte costituzionale.

che delle aziende che devono 177 milioni allo Stato possono risolvere il loro problema versando il 5 per cento

che queste stesse aziende hanno fatto (assolutamente in chiaro, per carità) donazioni significative a una delle forze che compongono la maggioranza di Governo, cioè alla

della Lega, se fossimo i 5 Stelle, diremmo che siamo di fronte al voto di scambio, a un traffico di influenze. Noi non diciamo questo;

a una brutta pagina che pagano i cittadini, in cui questo Governo si presenta come amico di alcuni e non certo come amico del popolo.

una breve replica, perché è curioso ascoltare chi ha ucciso il mercato delle sigarette elettroniche in Italia con una tassazione assurda, che ha colpito aziende innovative che avevano creato un mercato in grande espansione qualche anno fa. Lo stato di oppressione fiscale che il PD ha instaurato in Italia e che sta difendendo con questi interventi ha praticamente messo in ginocchio un intero settore. settore. Noi pensiamo che sia giusto procedere a una misura che metta in condizione quelle imprese e questo settore di poter respirare e di potersi liberare da un'oppressione fiscale assolutamente ingiustificata.

svolte all'estero che intendete regolarizzare dal punto di vista formale, noi chiediamo di escludere dalle irregolarità formali in particolare l'imposta sul valore aggiunto.

per essere tranquillo dal punto di vista ovviamente solo delle irregolarità formali? Chi è quel contribuente che, anche se ritiene di essere a posto, non pagherà questa nuova tassa? Ed è così vero che è una nuova tassa, che la somma di quello che prevedete di introitare nel 2019 e nel 2020 è il doppio di quello che prevedete di introitare con la somma di tutti gli articoli riferiti al decreto: 1,3 miliardi solo solo per questo articolo, mentre circa 600 milioni per la somma di tutti gli articoli. Altro che favore per le irregolarità formali! una vera e propria tassa su tutti i contribuenti: su quelli furbi, che premiate in altre occasioni, e su quelli onesti, che obbligate nel particolare a versare. Quindi, da una parte premiate coloro che non si sono comportati bene e dall'altra imponete agli onesti di pagare questa nuova imposta per soddisfare le vostre esigenze, che non sono quelle di migliorare il contrasto all'evasione fiscale e all'elusione, bensì di favorirle con gli altri articoli che sono previsti nel decreto-legge.

con il subemendamento 9.10000/11 proponiamo di stabilizzare, almeno per tre anni, il cosiddetto *bonus* bebè, altrimenti le famiglie non possono fare affidamento neanche su questo piccolo, quasi simbolico, aiuto che si dà loro. Le famiglie che oggi hanno figli ricevono dal fisco agevolazioni molto inferiori all'IVA che pagano in più, rispetto agli altri contribuenti, su tutti i prodotti che devono acquistare per i bambini. Chiediamo almeno che questo *bonus*, del tutto insufficiente, ma che è meglio di niente, sia pianificato per

regolari con il tentativo di dar loro la possibilità di chiudere ogni eventuale svarione che ci fosse stato nella loro amministrazione. Il Governo ha ritenuto di cedere a coloro che non volevano assolutamente andare incontro

piccolo pizzo per chiudere le irregolarità formali, perché la transazione sulle irregolarità formali, è il pizzo che l'amministrazione finanziaria impone ai contribuenti onesti, dato che se non fossero onesti, non commetterebbero irregolarità formali. FI-BP)*. La cifra può essere certamente ingente; è modica per l'unità, ma il numero delle imprese è tale che invoglia a chiudere la questione.

nei diversi temi che tratta, dalle nomine dei commissari ad altre questioni. Ecco perché noi ci asterremo su questo emendamento.

Presidente, abbiamo fatto presente anche in Commissione che questi sono i veri provvedimenti che si dovrebbero trovare in un decreto fiscale, cioè delle misure che mirano a ripristinare un giusto rapporto

Signor Presidente, intervengo perché l'emendamento 9.0.4 riguarda un tema di equità e di giustizia nei confronti di tutti i contribuenti e i cittadini. Noi, con questo emendamento, chiedevamo alla maggioranza di permettere al cittadino contribuente, che si avvale della cosiddetta pacificazione fiscale o di quello che ne è rimasto, di poter utilizzare in pagamento i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. La riterremmo una misura di giustizia e di rispetto verso il cittadino, che quando non paga viene vessato dallo Stato e quando, invece, ha dei crediti nei suoi confronti, non può neppure utilizzarli.

si sono sempre rivolti al popolo e hanno sempre richiamato l'onestà, per dire di votare a favore di una richiesta che vuole giustizia ed equità: permettiamo di pagare con i crediti verso lo Stato.

ho scritto un disegno di legge, poi trasformato in emendamento, proprio prendendo spunto da una vicenda che a voi della maggioranza dovrebbe essere molto nota. Mi riferisco all'imprenditore Bramini,

voleva far sì che ci fosse da questo momento in poi una compensazione tra crediti e debiti. Ora vi mettiamo alla prova e vedremo, secondo me, anche in questo caso quanto questo Governo giallo-rosso sia bravo a parlare, ma molto cattivo ad agire. *(Applausi

intervengo sull'articolo 10, quindi su un articolo che riguarda in particolare la fatturazione elettronica. Si tratta di un tema che a noi di Fratelli d'Italia è particolarmente caro, caro, perché va a gravare pesantemente su quella piccola e media impresa che è il cuore pulsante della nostra economia. Voi, cari amici della maggioranza, avete previsto oltre un miliardo di gettito per le casse dello Stato, attingendo appunto alla fatturazione elettronica. Fermo restando che io ne dubito molto e che sarò lieto di aspettarvi, tra dodici o quindici mesi, per fare i conti e vedere se effettivamente avrete introitato questo denaro, anche ammesso che ciò accada (e, ripeto, ne dubito fortemente), questo denaro viene preso dai poveri imprenditori e artigiani, per essere indirizzato all'assistenzialismo. Cioè vogliamo investire sull'assistenzialismo, facendone pagare l'onere alle piccole imprese del nostro Paese. Quelle piccole imprese che già si trovano a competere in un mercato difficile, con uno Stato che non gli dà una libertà economica vera. Ecco, questa è fondamentalmente la fattura elettronica: fare cassa sulle spalle di chi lavora, per introitare quei soldi e girarli a chi non lavora e magari ha ben poca voglia di lavorare. senatore Damiani dell'articolo 10. In quest'Aula ne abbiamo già discusso qualche giorno fa e anche noi interveniamo, oggi, per esprimere il nostro forte disappunto

che ci chiedono non di ritardare, ma di posticipare l'entrata in vigore della fatturazione elettronica di un solo anno. anno. La proposta che abbiamo lanciato in quest'Aula e nelle Commissioni è stata purtroppo bocciata da un'alleanza politica molto strana, che vede il Governo unito al Partito Democratico nel pensare a questa riforma. Noi esprimiamo il nostro disappunto, perché ce lo chiedono i cittadini in questo momento particolare. richiesta anche in virtù del fatto che oggi abbiamo ancora delle grandi difficoltà nel nostro Paese: una grande parte del nostro territorio ancora oggi viaggia con il 2G, mi dovete spiegare, allora, come fa a partire una fattura elettronica, se il sistema è ancora quello del 2G.

a regime il sistema di interscambio e non realizzi la banda larga su tutto il territorio nazionale. Come si può chiedere ai contribuenti - soprattutto a quelli piccoli - di assumersi i costi che lo Stato sta invece scaricando su di loro? Questa è davvero

nella direzione della spina dorsale portante di questo Paese.

Quindi, sostenere che questo Governo non si sia occupato del tema non è la verità. Poi si poteva fare di più: è sempre così. Quando si è all'opposizione,

che il Governo poteva fare. Siamo intervenuti in questa direzione, sicuramente rivolgendo l'attenzione a tutti gli artigiani, agli imprenditori e alle piccole e medie imprese che chiedevano un segnale da parte dell'Esecutivo e ciò deve essere riconosciuto in quest'Aula. Senatore La Russa, Signor Presidente, ha ragione il Capogruppo della Lega: quando si è all'opposizione, si è più liberi di dire le cose che si pensano. Il nostro problema è proprio questo: abbiamo l'impressione che la Lega vorrebbe, ma non può.

adesso non è tanto di essere al Governo, perché sentir dire che non possiamo contraddire in Europa quello che ha fatto il Governo di sinistra mi pare un po' troppo, anche perché - grazie a Dio

silenzio che la Lega debba accettare di cambiare la propria opinione, e non perché è al Governo e ha rispetto del bilancio, ma perché l'altra parte

noi abbiamo cercato di trovare ogni soluzione per fare in modo che la fattura elettronica non si applicasse. Abbiamo chiesto la soppressione, abbiamo chiesto la dilazione temporale e poi abbiamo anche chiesto, con questo emendamento, di applicarla al di sopra di un fatturato minimo.

economica del nostro Paese. Le piccole e medie imprese sono quelle il cui fatturato si aggira intorno ai 500.000, 700.000 o 800.000 euro. Un esercizio "Sali e Tabacchi" oggi non è più quello che vende il chilo di sale, ma è quello che fattura almeno 600.000 euro all'anno per la vendita dei Gratta e Vinci: è la più piccola impresa italiana. Allora, io comprendo l'accorato appello del Presidente del Gruppo Lega, il senatore Romeo. Lo capisco perfettamente, perché deve dare

gli investimenti, che avremmo fatto in modo che nella prima finanziaria del primo Governo di centrodestra ci sarebbe stato un abbattimento importante della pressione fiscale, sia nazionale che locale.

portata avanti dal Governo di centrosinistra, dal Governo Gentiloni Silveri, cancellandola, si stanno giustificando con chi li ha votati, con chi ci ha votato, con chi ci ha sostenuto, dicendo che tutto ciò non si può fare. Allora, qual è la motivazione che costringe i nostri amici della Lega a restare in un Governo che, anziché andare nella direzione di aiuto alle imprese e allo sviluppo del nostro territorio, serve soltanto per mantenere una posizione di Governo e di potere all'interno di questo Parlamento e all'interno di una situazione così difficile? Ma fanno bene i colleghi del MoVimento 5 Stelle a farsi due risate sotto i baffi, perché in questo caso la componente di centrodestra di questo Governo è annichilita, quasi scomparsa, e quasi svanita, in particolare sulla questione del decreto fiscale, delle tasse e della manovra di bilancio, che doveva essere un rilancio dell'attività e delle piccole e medie imprese di questo Paese.

esitato un solo istante: avremmo difeso l'economia e avremmo abbandonato il Governo. E questo chiediamo ai nostri amici della Lega: lasciateli andare alla deriva e rimaniamo fermi sugli impegni presi con gli elettori il 4 marzo.

di una storia lunga, Presidente; una storia che vede una vessazione continua negli ultimi anni - con l'eccezione parziale dei periodi in cui governava il centrodestra - a danno dei lavoratori autonomi. C'è un un modo di immaginare i rapporti sempre di sospetto nei confronti dei lavoratori autonomi, e quindi, in questo caso, di coloro che sono chiamati alla fatturazione elettronica o delle piccole aziende. L'emendamento 10.100 (testo 2)/2, che assomiglia a uno più complesso, ma simile, di Fratelli d'Italia, presentato dal senatore De Bertoldi, ci dà l'opportunità di ricordare agli amici della Lega che questa impostazione culturale si è vista anche oggi. Sapete qual è la riprova?

imprese, per gli artigiani e i commercianti sono stati bocciati non solo con il voto - già sufficiente - dei partiti di Governo, ma anche con il voto compatto di tutta la sinistra; coerente, per carità, con la sua lunga storia di vessazione nei confronti delle piccole e medie aziende, nei confronti degli artigiani e dei commercianti. Non siete in buona compagnia.

Signor Presidente, vorrei aggiungere qualcosa in relazione a quanto viene raccontato come un disastro, ovvero la fatturazione elettronica. Iniziata questa discussione ho acceso il mio tablet - cinque minuti fa - e ho attivato la fatturazione elettronica per la mia azienda. Ebbene, il costo annuale di tale attività sarà di 35 euro; quindi, tutta la difficoltà di cui parlate per una piccola e media azienda come la mia - e come tante altre piccole e medie aziende italiane - non esiste. Probabilmente, chi parla da tempo ha perso il contatto con la realtà, da tempo non gestisce più autonomamente le proprie aziende. M5S)*. Capisco che ci sono categorie che hanno maggiori difficoltà nell'utilizzo degli strumenti elettronici, ma per loro c'è sempre lo studio del commercialista che, almeno nelle mie zone, per una piccola cifra

star salvando la gente, perché salvate solo imprese piccolissime, come ha detto il senatore Mallegni. Le imprese vere sono quelle che fatturano molto di più, per guadagni di più, per guadagni certamente limitati, non certo da 6.000 euro al mese, ma molto inferiori. Invece, a persone che di fatto incasseranno dai 1.500 ai 2.000 al mese di guadagno

si spendono decine di minuti per poche fatture, magari per pochi euro. Questa è la situazione reale. Questo è il Paese reale. Bisognerebbe capirlo e non soltanto dire di rappresentarlo.

stiamo uccidendo la piccola e media impresa italiana: oggi purtroppo certificherà questo la votazione che faremo. I nostri colleghi della Lega e del Movimento 5 Stelle ogni tanto ci danno qualche spunto, come ad esempio il wi-fi; sì, è bellissimo usare il wi-fi del Senato, ma vorrei sapere come si fa a spedire una fattura elettronica con il 2G, che troviamo tranquillamente nei Comuni più piccoli. Dicono che non si può prorogare la fatturazione elettronica perché è colpa del Governo Gentiloni Silveri, ma il reddito di cittadinanza è colpa del Governo 5 Stelle, e non del Governo Gentiloni Silveri. Se dobbiamo trovare 2 miliardi di euro per prorogare di un anno la fatturazione elettronica e dare respiro a chi lavora, possiamo tranquillamente ridurre il reddito di cittadinanza. È inammissibile dare reddito a chi non lavora, a chi è un nullafacente, a chi proprio non fa nulla per il nostro Paese. Noi chiediamo solo aiuto per le nostre piccole e medie imprese, che sono sempre state quelle che hanno portato avanti l'Italia,

i nostri amici della Lega possano permettere una cosa del genere. Quelli sono i nostri elettori, coloro che ci hanno sempre votato, il popolo delle partite IVA, che voi state scambiando con il popolo dei fannulloni.

Signor Presidente, noi mai avremmo pensato che la trattazione della fattura elettronica determinasse un dibattito tra la coalizione che fu di centrodestra così animato e così appassionato. Sinceramente a noi non interessa molto il il rispetto più o meno acclarato del vostro programma. Non vi dovete tanto fare domande circa il giudizio sulla fatturazione elettronica e sulle vostre valutazioni intorno a questo tema; piuttosto dovreste chiedervi come mai le vostre promesse elettorali, quelle del centrodestra, di una *flat tax* che era alle porte, sono diventate nuvole, sono svanite nel nulla e credo che mai vedremo la famosa *flat tax* nel nostro Paese. Magari interrogatevi su questo e non aprite una diatriba tra voi sulla fatturazione elettronica, che pure è un tema

perché non nasce oggi, cominci ad entrare a regime e faccia parte della normale gestione del fisco del nostro Paese. Prima il relatore di minoranza ha parlato della fatturazione elettronica come infrastruttura del nostro sistema fiscale. Io credo che e non lo dico io, non lo dice il Partito Democratico, ma lo dicono la Corte dei conti e il Ministero delle finanze - la tracciabilità sia un valore aggiunto per poter portare innanzi una lotta all'evasione più credibile. Noi abbiamo un'evasione IVA di 36 miliardi l'anno, è un primato europeo: è un'evasione del 13 per cento superiore alla media europea e qualche domanda ci dobbiamo porre. Non credo che tutti siano evasori, e non lo crede il Partito Democratico, ma la tracciabilità è

c'è un adeguamento tecnologico di cui si deve tener conto, e in termini non tanto di costi, ma di tempi necessari per farlo. Su quello non siamo pregiudizialmente contrari, ma pensiamo che questa azione dilatoria

per un fisco equo. In questi anni le nostre riforme hanno consentito un abbassamento, seppur non altissimo, della pressione fiscale, nonché un recupero importante di evasione fiscale. Non lo dico io, ma lo dice l'Agenzia delle entrate: 20 miliardi di recupero, più 5,8 rispetto all'anno precedente. Analogamente, sono stati riscossi molti più ruoli rispetto agli anni passati, e sempre l'Agenzia delle entrate in Commissione finanze ci ha esplicitato questi risultati: 12 miliardi rispetto agli 8,8 miliardi dell'anno precedente. noi non siamo per lo Stato fiscale, ma siamo per uno Stato in cui le tasse si paghino per quello che è giusto pagare e, quindi, per far sì, una volta che avvenga questo, che si abbassi conseguentemente anche la pressione fiscale.

devo segnalare un refuso, perché il periodo aggiunto all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 2015 in realtà è aggiuntivo e non sostitutivo. Posso leggere l'intero emendamento, se necessario.

"Per il periodo di conservazione gratuita delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il *partner* tecnologico Sogei SpA non può avvalersi di soggetti terzi."».

Signor Presidente, come è stato sottolineato in precedenza, noi contestiamo questo modo di procedere, in particolare della 5ª Commissione.

della Lega e del MoVimento 5 Stelle, dovesse essere concluso. *(Applausi della senatrice Lonardo).* Oggi, invece, abbiamo avuto più rinvii e più pause, perché evidentemente non erano pronti. Se non erano però pronti, signor Presidente, noi avevamo deciso che la Commissione avrebbe lavorato sabato e domenica. Come mai questo non è successo? Non credo che si possano considerare le istituzioni come qualcosa con cui lavarsii piedi*.* È inaccettabile! *(Applausi dai Gruppi

FI-BP).* Per favore, assumiamo un atteggiamento responsabile, idoneo all'Istituzione e al provvedimento del quale stiamo discutendo.

tempistica dei lavori della Commissione. Capisco e mi auguro che prossimamente, per quanto riguarderà gli altri provvedimenti, si tenga conto di quanto viene stabilito in Conferenza

FI-BP)*. Presidente, spezzo una lancia in favore del Presidente della 5a Commissione (i membri della Commissione ne saranno sorpresi). Il problema che qui abbiamo

per dare la possibilità all'Assemblea di poter verificare l'emendamento, possiamo anche accantonarlo, non succede nulla, in modo che ognuno di voi abbia la possibilità di poterlo leggere e verificare la compatibilità della prima

perché il Governo e la maggioranza non erano pronti. È la dimostrazione per cui oggi siamo a questo emendamento, che si può accantonare, Presidente; il problema però c'è stata una dialettica nella maggioranza su diversi emendamenti che si è scaricata sulla funzionalità della 5a Commissione. È questa, Presidente, la questione su cui lei deve

Presidente, con tutti gli sforzi di benevolenza, quella che lei chiama modifica formale è una modifica sostanziale e se non fosse stato per l'intervento dei colleghi dell'opposizione, noi avremmo votato

troppo in prossimità dei lavori dell'Assemblea, viene utilizzata dalla maggioranza come tagliola per fare in modo che i provvedimenti, gli emendamenti e le proposte suscettibili di creare imbarazzo nella maggioranza non possano arrivare al voto. *(Applausi dai Gruppi FdI e PD)*. Questo non è accettabile, Presidente. Ancora una volta le chiediamo di fare da garanzia soprattutto e principalmente per le opposizioni perché la maggioranza, ripeto ancora, si difende da sé perché il Governo è forte e ha dalla sua parte i numeri che fanno la differenza.

senatore Marcucci

quindi che ci debba essere attenzione nei confronti delle procedure e non penso che si debba accantonare. Credo che il relatore debba avere il coraggio di dire che, evidentemente, non sa fare il proprio mestiere e che debba presentare un suo nuovo emendamento, sostitutivo di questo. Così si dovrebbe fare.

Signor Presidente, ricevere una critica da un Gruppo parlamentare a cui nella scorsa legislatura sono state bocciate delle leggi in Corte costituzionale

Adesso sono chiare due cose: che il clima si sta deteriorando e, soprattutto, che alle ore 21 noi non chiuderemo questo provvedimento, e non certo per colpa delle opposizioni. Semmai

visto che sono le 20,10, rinviare a domani mattina la prosecuzione dei lavori.

Rapidissimamente volevo avvisare il collega La Russa che questa sera gioca la Juve, mentre l'Inter gioca domani sera. Quindi possiamo andare avanti.

possibile. Se lei ha da dire qualcosa, lo dirà poi alla fine dei lavori di questa serata.

Siccome qui c'è un problema che riguarda l'interpretazione dell'emendamento 10.20 nella riformulazione proposta dal relatore, emendamento sia accantonato, in modo da dare la possibilità a tutti di rileggerlo e di leggere anche gli emendamenti successivi, ove

si impone allora l'obbligo della fatturazione elettronica, ma almeno si voglia sgravare l'obbligo da parte del contribuente di archiviare la documentazione informatica una volta inviata alla pubblica amministrazione o agli enti preposti.

Dobbiamo essere vicini al contribuente e ai cittadini e non dobbiamo continuamente contribuire con queste imposizioni che sono gravose e onerose.

si sia occupato di amministrazione sa che una disposizione di questo genere non ha senso. Il diritto alla detrazione va esercitato entro un termine e non è assolutamente ammissibile che le fatture ricevute nel mese di dicembre o comunque a fine anno debbano avere un trattamento diverso rispetto a tutte le altre. Quindi, noi abbiamo proposto - ma non siamo i soli, anche

sono volti ad aumentare la detrazione - almeno per le persone che hanno superato i sessant'anni - per tutto ciò che riguarda le spese di farmaci veterinari. In un momento in cui la sostenibilità del nostro sistema sanitario è messa a dura prova, sappiamo perfettamente come per una persona anziana prendersi cura di un animale, oltre ad ad aiutare la promozione dello stile di vita per una vecchiaia in salute, permette anche di non cadere in depressione. in depressione. La mancanza di attività fisica e la solitudine di un anziano possono essere sicuramente migliorate dalla presenza di un animale. Sappiamo perfettamente che, se non si possono detrarre le spese veterinarie, gli anziani arrivano persino a togliere il cibo dalle loro tavole per poter curare il loro animale da compagnia. Quindi, chiedo veramente una sensibilità all'Assemblea

randagismo nel Centro-Sud - se le persone fossero incentivate ad adottare, ad esempio, un cane o un gatto nei canili o nei gattili, che invece sono a spese dei Comuni e quindi dei cittadini.

le fatture emesse verso soggetti esteri perché l'Italia, come sappiamo tutti, farà da pilota a livello europeo rispetto all'entrata in vigore anticipata della fatturazione elettronica. quindi necessario per i soggetti che emettono fatture verso l'estero avere un riscontro di tali fatture da parte dello Stato. Questo è il quadro generale.

e che comunque rappresentano i contribuenti presso l'Agenzia delle entrate e le commissioni tributarie, la famosa posta elettronica certificata (PEC) per ricevere comunicazioni tramite questo tipo di modalità.

la questione delle detrazioni per le spese veterinarie, ferme da moltissimo tempo e che incidono molto relativamente (perché il massimo della detrazione è di fatto pari a circa 50 euro, quindi una somma abbastanza piccola),

non so se mi sta ascoltando - a tenere in considerazione questi emendamenti, così come quelli successivi che abbiamo presentato anche trasversalmente, che riguardano sia la questione dell'IVA

degli anziani). Oggi queste detrazioni sono davvero irrisorie: pensate, non arrivano neanche a 130 euro. È un'assurdità se si pensa che le spese veterinarie in Italia sono davvero troppo onerose; per non parlare di quelle dei farmaci dedicati agli animali. Ebbene, queste spese veterinarie sono talmente alte che spesso, purtroppo, diventano anche causa di abbandono del proprio animale domestico,

nell'utilità di aumentare le detrazioni fiscali per le spese veterinarie a favore delle persone più anziane. La comunità scientifica internazionale ha riconosciuto la validità della *pet therapy*, cioè della terapia fatta con l'utilizzo degli animali domestici a favore di bambini che hanno patologie gravissime, a favore di disabili e di persone che hanno problemi psicologici, problemi mentali, di depressione. Questo può essere davvero un investimento per i

Signor Presidente, colleghi, anch'io rivolgo un appello al relatore e al rappresentante del Governo nella speranza che voglia accogliere questi emendamenti, sui quali non spendo ulteriori parole, perché mi associo a quanto già detto dalle colleghe De Petris e Giammanco che con me

Ricordo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che l'aspetto relativo all'ambiente e agli animali è parte fondante del loro programma

stanno seguendo le indicazioni già seguite da tempo dalle amministrazioni comunali a guida di molti sindaci del centrosinistra. Ricordo a tutti quello che è stato fatto anni nel Comune di Roma, quando con le giunte di centrosinistra fondammo l'Ufficio diritti animali che divenne elemento di traino per altre amministrazioni. Ha detto molto bene la collega Giammanco: in tante famiglie, in particolare di anziani, le spese veterinarie sono una voce importante, lì dove, davanti a una solitudine, per mille ragioni sociali che non è il caso di approfondire in questo momento, un amico non umano, un figliolo a quattro zampe, diventa il centro della vita e della solitudine di questi anziani. Ci sono anziani che hanno anche due, tre o quattro animali in casa e che spesso si privano, si privano, loro stessi, di somme di denaro per curare i loro animali. Un altro dato importante - ed è stato sottolineato bene il tentativo di ridurre l'IVA sul cibo e sui medicinali veterinari. Non possiamo pensare che il cibo per cani e per gatti, per piccoli roditori, per uccellini e per tutti gli animali che sono nelle nostre case sia sia tassato come bene di lusso. Avere un animale in casa, molto spesso salvato da un canile, molto spesso raccolto dalla strada, non è certamente un'ostentazione del lusso. Proprio per questo

Mi piace ricordare che Alzheimer, autismo e disabilità sono tutte problematiche che prevedono l'utilizzo degli animali per la terapia, che sta dando fortissimi risultati. Fra le tante, una delle ultime sperimentazioni progettuali che si sta facendo sul territorio prevede l'adozione di cani tripodi, quindi con disabilità, da accostare in programmi di *pet therapy*, per dimostrare ai ragazzi giovani che la disabilità è superabile. poiché credo che non comprometterebbe i conti dello Stato approvare questa proposta, inviterei il relatore e il Governo a riprendere in considerazione l'approvazione di questi emendamenti.

Presidente, sono piuttosto perplessa. Infatti, anche dalle dichiarazioni dei colleghi si capisce quanto limitato sarebbe il costo per lo Stato. Non solo: avevo anche trovato la copertura per queste spese minime per il bilancio dello Stato, ma importanti per le famiglie,

sapendo che sarà solo di un anno, voterò a favore del mio emendamento, che chiede la detrazione per le spese che le famiglie sostengono per l'iscrizione in palestra dei propri ragazzi o per le persone anziane. Credo che ciò rientri sempre in un progetto di sanità pubblica e di prevenzione e, per quanto riguarda i ragazzi, investa anche la loro educazione,

anche intellettualmente (perché una palestra per l'anziano significa anche coordinamento e mantenere vigile il proprio sistema di riflessi). Spero che l'Assemblea Spero che l'Assemblea risponda, almeno su questo, positivamente. Si tratta di salute pubblica, non di favorire qualcuno. È inutile esaltarsi per un anno di proroga del *bonus* bebè, quando non si aiuta la famiglia a crescere i propri figli in modo salutare.

che c'è un lavoro in corso svolto in parte in Commissione finanze, ma anche in altri luoghi della tecnica, del diritto e dell'elaborazione urbanistica, possiamo trasformare l'emendamento in ordine del giorno perché abbiamo costruito in Commissione un'adeguatezza di interesse.

ne abbiamo discusso in Commissione e saremmo d'accordo per la trasformazione in ordine del giorno. Riteniamo che, come nel mille proroghe di luglio sia stato abrogato lo *split payment* per i professionisti, così dal 1° gennaio 2019 debba essere abrogato questo strumento antielusivo vista l'entrata in vigore della fatturazione elettronica, che questo Governo interpreta non come un provvedimento di progresso sociale, ma come uno strumento antielusivo. Sarebbe una duplicazione a ulteriore aggravio dei contribuenti.

nelle more di una sentenza del Consiglio di Stato, di definire le autorizzazioni e chi le deve concedere per poter consentire a tutte le aziende che si occupano di riciclo e di economia circolare di poter continuare a lavorare perché ormai gli impianti sono fermi. So che siamo diventati un disco rotto però, per cortesia, per però, per cortesia, per un Governo, che pomposamente si definisce Governo dell'economia circolare, che fa convegni su convegni e che parla di *green economy*, di rifiuti e di tutta una serie di iniziative che vanno nell'ordine di idee che le aziende debbono lavorare per la sostenibilità ambientale, mi sembra veramente un paradosso. Non è una questione di interessi di parte perché su tale questione si sono mossi tutti, da Legambiente fino a Confindustria, passando per tutte le associazioni. Stasera l'emendamento sicuramente sarà respinto perché ho visto i pareri del Governo, però lo ricorderò tutte le volte che vi definirete Governo dell'economia circolare.

B)*. Comunico che è stato riproposto all'Assemblea un emendamento del relatore in materia di concessioni autostradali, già presentato in Commissione e giudicato ammissibile dal Presidente del Senato. Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per le ore 21,30.

io credo che quello che abbiamo detto finora non sia servito evidentemente a niente. Il Governo presenta un emendamento sulle concessioni autostradali

noi non abbiamo visto l'emendamento. Sono le 21,05. L'emendamento dovrebbe, evidentemente, ritornare in Commissione. Abbiamo visto troppe cose in quest'Aula oggi per pensare

Colleghi, c'è un limite a tutto. Questo no! Veramente, questo no! La Commissione abbia la dignità di riunirsi e di produrre in maniera trasparente un emendamento, che noi ora non abbiamo neanche testualmente! Ci sono emendamenti fantasma che girano in quest'Aula. Non lo possiamo permettere. Si riunisca la Commissione e non si diano termini per i subemendamenti! Non abbiamo materiale per emendare, signor Presidente! Manca l'emendamento.

che, erroneamente, è stato ritirato. Ci siamo accorti solo adesso che è lo stesso, uguale e identico. Sono d'accordo sul fatto di dare il tempo necessario agli uffici per poter presentare, eventualmente, subemendamenti. Comprendo anch'io sia un termine troppo ristretto. Quindi, siamo disponibili a rinviarlo. Però, è un emendamento identico. Arriva adesso perché ci siamo accorti che, in modo sbagliato, è stato ritirato in Commissione. Chi ha fatto parte della Commissione finanze, e qui vi sono degli illustri membri commissari, sia del Partito Democratico

tentativo dell'ultimo minuto di far rientrare qualcosa. Solo questa è la motivazione. Quindi, se la Presidenza e i Gruppi sono d'accordo, diamo più tempo per la presentazione di eventuali subemendamenti, ma non creiamo un caso che, sinceramente, non esiste.

Signor Presidente, le confermo che, preso atto delle giuste richieste delle nostre costruttive opposizioni, domani convocheremo la 6a Commissione alle ore 9

le espressioni di solidarietà e vicinanza al territorio del Basso Salento sul quale, per diversi giorni, si è accanita un'ondata di maltempo particolarmente violenta, culminata l'altro ieri con un vero e proprio tornado che ha spazzato via oltre 20 chilometri di costa nel Capo di Leuca. È stato un fenomeno di una violenza distruttiva senza precedenti, riconosciuto come un F2 che ha sprigionato venti a oltre 200 chilometri orari, facendo crollare chiese, isolati, tante abitazioni; ha distrutto diverse strutture turistico-ricettive, insediamenti produttivi, non solo agricoli, affondato decine e decine di imbarcazioni, messo in ginocchio la circolazione dei convogli dei trasporti pubblici locali e intere comunità cittadine. Solo un vero e proprio miracolo non ci fa aggiungere oggi a tutto questo l'elenco di vittime, perché, solo per circostanze fortuite, non ci sono state vittime. vittime. Con questo mio intervento oggi qui in Aula desidero innanzitutto ringraziare i sindaci dei Comuni interessati, come Tricase, Patù e Morciano, ed il presidente della Provincia di Lecce, che hanno da subito avviato la macchina dei soccorsi e di protezione civile e in tempo da record messo in piedi un tavolo per gestire l'emergenza. In questa sede, però, desidero anche ribadire la mia disponibilità ad essere portatore delle istanze di necessità di questo territorio e, soprattutto, chiedere a quest'Assemblea, a lei, signor Presidente, e soprattutto al Governo (che è già scappato via) di prestare massima attenzione alle istanze che perverranno. Il Salento è forte, ha tempra dura e si alzerà in fretta, è vero, ma abbiamo anche bisogno che il Governo e il Parlamento diano segnali di vicinanza.